piedi).* Purtroppo anche oggi, 25 giugno, abbiamo un altro lutto sul lavoro: si tratta di Giovanni Terrana, un operaio di sessantacinque anni, morto questa mattina a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, cadendo da una impalcatura di circa bene, purtroppo non è l'unica vittima di incidenti sul lavoro che si susseguono con una allarmante e inaccettabile frequenza. Solo negli ultimi giorni,

che è morto quando la gru accanto a cui lavorava è caduta e col suo lungo braccio lo ha colpito mortalmente.

il 21 - quindi vedete la frequenza è incredibile - Valerio Salvatore, giovane romano di appena ventinove anni, è caduto dal tetto di un'azienda a Campoleone, in provincia di Latina, da circa dieci metri e non ha avuto scampo. Mirko Schirolli il 21 giugno, nella stessa giornata, è morto in una fabbrica in provincia di Mantova, schiacciato da un macchinario industriale. Come vedete, è un bollettino di guerra incredibile. Il giorno prima, il 20 giugno, Pierpaolo Bodini, di diciotto è morto per il crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all'interno di una cascina a Brembio, in Lombardia, nel lodigiano. Queste vicende

dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola. È un bollettino allarmante, incredibile e inaccettabile, che tutte le forze politiche hanno sottolineato, che il Presidente della Repubblica ha messo al centro di un suo specifico intervento e che noi non possiamo ignorare. In accordo con il Presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro si stanno intensificando i lavori della Commissione per portare una relazione all'Assemblea, ma dalle parole bisognerà passare ai fatti, e cioè alla normativa. Credo Credo però che, al di là della normativa, una presa di coscienza, una consapevolezza della centralità di tale questione debba attraversare tutte le forze politiche e portarci a risposte le più urgenti possibili, perché il bollettino di vera e propria guerra non abbia a proseguire Grazie a tutti.

finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto

al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio. Nella seduta di oggi, senza orario di chiusura, si svolgerà la discussione generale del decreto-legge coesione. Dopo la preannunciata posizione della questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione bilancio, si proseguirà con la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sul Terzo settore, già approvato dalla Camera dei deputati. Le dichiarazioni di voto e la chiama sulla fiducia sul decreto avranno luogo domani, a partire dalle ore 10. Resta confermata, per la seduta di domani, alle ore 15, la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno La consegna del testo delle Comunicazioni rese alla Camera dei deputati avrà luogo nel corso della mattinata. Il calendario dei lavori della settimana corrente è altresì integrato con la discussione del disegno di legge concernente la delega al Governo in materia di florovivaismo, per il quale la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per complessive tre ore, escluse le dichiarazioni di voto. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani. Il calendario prevede inoltre il decreto-legge sulle rappresentanze sindacali militari, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ove trasmesso in tempo utile. Giovedì 27 giugno, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della difesa, dell'agricoltura e dell'università. Nelle settimane successive, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i seguenti decreti-legge: agricoltura e imprese di interesse strategico, nella settimana dal 2 al 4 luglio; liste di attesa, liste di attesa, nella settimana dal 9 all'11 luglio; protezione civile e semplificazione edilizia e urbanistica, nella settimana dal 16 al 18 luglio; sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, nella settimana dal 23 al 25 luglio. luglio. Giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio, alle ore 15, avrà luogo il *question time*. Su richiesta di un Gruppo parlamentare, la Conferenza dei Capigruppo altresì convenuto di inserire nel calendario dei lavori, a partire da martedì 17 settembre, la discussione del disegno di legge, sottoscritto da un terzo dei senatori, concernente disposizioni in materia di morte medicalmente assistita. È stato infine stabilito di riassegnare in sede deliberante i seguenti disegni di legge, già conclusi in sede redigente: nuova denominazione Giornata vittime dei disastri ambientali, istituzione del Museo del Ricordo, promozione delle manifestazioni in abiti storici, centenario della Fondazione della città di Latina.

tra maggioranza e opposizione, tant'è vero che non c'è stato alcun problema per quanto riguarda i vari lavori che si sono svolti durante la discussione degli emendamenti. emendamenti. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del PNRR. Permettetemi di ringraziare il presidente della Commissione Calandrini, che ha guidato con grande piglio e con serenità - come dicevo prima - un lavoro che è stato svolto in modo sereno da entrambe le parti. Ringrazio altresì il sottosegretario Siracusano, che è stato sempre presente nelle varie discussioni, e soprattutto il ministro Fitto, che

113 miliardi di euro. E ciò permette all'Italia di essere il Paese che più sta lavorando e producendo in termini di PNRR.

nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione nei settori strategici: risorse idriche, infrastrutture per il rischio geologico e protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese

L'articolo 3 configura la cabina di regia per il Fondo di sviluppo e coesione e il confronto tra Stato, Regioni e Province autonome per il coordinamento, la complementarità, la sinergia e il monitoraggio. All'articolo 4 ci sono le disposizioni per l'individuazione da parte delle amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, con un elenco di interventi prioritari nei settori strategici. Al comma 7 dell'articolo 4 c'è il piano strategico per la ZES unica del Mezzogiorno. All'articolo 5 ci sono disposizioni di monitoraggio e rafforzamento degli interventi prioritari, con relazioni semestrali. 6 troviamo il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. I commi 5 e 6 dell'articolo 6 prevedono la convenzione con la società *in house* Eutalia Srl per l'attuazione di specifiche progettualità. L'articolo 7 definisce la premialità per le Regioni e Province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici. L'articolo 8 reca le norme di finalizzazione ad attivare gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa e per il fondo per una transizione giusta. L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione, con funzioni di controllo e di autorità di *audit*, sia composto da cinque unità. con delibera CIPESS, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione anche a quelle Regioni con cui non sia stato sottoscritto l'Accordo per la coesione. L'articolo 11 interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. per cento la quota di risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni devono destinare al Mezzogiorno. L'articolo 12 interviene sui contratti istituzionali di sviluppo per la ricognizione delle funzioni di responsabile unico del contratto e per la revisione della *governance*. L'articolo 13 dispone sulle zone logistiche semplificate, introducendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e di quelle nuove. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 aumentano la disponibilità del Fondo di sostegno per i Comuni marginali. L'articolo 14 tratta del risanamento del sito industriale di Bagnoli (provvedimento molto sentito). Il comma 4 dell'articolo 14 reca disposizioni per la valorizzazione energetica e la gestione dei rifiuti in Sicilia. L'articolo 15 reca norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai Comuni marginali. L'articolo 16 prevede specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale. L'articolo 17 disciplina l'autoimpiego nel Centro-Nord Italia per il sostegno di attività imprenditoriali e libero-professionali per gli *under* 35. L'articolo 18 disciplina le misure denominate Sud 2.0 per gli *under* 35 nel Mezzogiorno. L'articolo 19 prevede che il Ministro del lavoro si avvalga di soggetti gestori delle misure per l'autoimpiego nel Centro-Nord e Sud 2.0. Lascio ora la parola alla collega Murelli.

dall'articolo 20 al 29, nel decreto coesione, ci sono misure per il mercato del lavoro, in particolare per rafforzare l'occupazione delle categorie dei lavoratori più svantaggiate in generale del Mezzogiorno. A disposizione per la promozione dell'occupazione ci sono oltre 2,8 miliardi di euro, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-27 e sulle risorse della Misura 5 del PNRR, dedicata alle politiche attive collegate al programma GOL, a cui si aggiungono le risorse per la riconversione della competenza dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi. Le principali misure in materia di lavoro sono la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività di incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica; l'iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifica al funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Al fine di incrementare l'occupazione, il decreto coesione prevede inoltre tre esoneri contributivi per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni. Si tratta del *bonus* giovani, che consiste nell'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro per per l'assunzione di giovani di età non inferiore ai trentacinque anni; c'è il *bonus* donne, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro, senza applicazione dei limiti di età; la terza misura riguarda il *bonus* ZES, che sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno, attraverso uno sgravio contributivo del 100 per cento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nei limiti di 650 euro, per ciascun lavoratore assunto, per datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti. Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e coesione territoriale, quali, tra l'altro, la revisione della disciplina e il finanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale; la ricognizione dello stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo; l'estensione delle misure di semplificazione dei benefici fiscali previsti per le ZES uniche e anche per le zone logistiche semplificate; le misure volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio. Infine, sono introdotte misure specifiche in materia di istruzione, università e ricerca, con rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici, assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, e l'accelerazione di impiego delle risorse del Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027, destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive, dei laboratori tecnici e degli arredi negli asili; investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socioeconomico e abitativo, per il recupero dei siti industriali cultura, con l'approvazione del Piano di azione per il Programma nazionale cultura; sulla sicurezza, attribuendo a specifica operazione nel programma Sicurezza per la legalità 2021-2027 la qualifica di operazioni di importanza strategica. In aggiunta, ci sono gli emendamenti approvati in Commissione bilancio la scorsa settimana, che riguardano in particolare gli emendamenti dei relatori, che rimpolpano di 330 milioni la dote finanziaria assegnata dalla legge di bilancio per il 2024 ai contratti di sviluppo, i programmi straordinari di investimento, siglati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*; 80 milioni sono autorizzati per quest'anno, passando così da 190 ai 270 milioni; 250 milioni per il 2025, passando dai 310 ai 560 milioni. Il secondo emendamento riguarda i segretari comunali e provinciali. È aumentata È aumentata l'assunzione di 245 nuovi segretari generali comunali e provinciali. L'altra buona notizia riguarda gli enti locali: è stato approvato un emendamento che limita il vincolo di cassa alle entrate da trasferimenti mutui; via libera anche ai 18 milioni fino al 2029 per la metro M1 di Milano. Infine, grazie all'approvazione di un emendamento firmato da tutti i Capigruppo di tutte le forze politiche, i Comuni avranno più tempo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI fino al 2024. Anch'io vorrei concludere ringraziando direttamente la Commissione, i colleghi relatori, i funzionari, la sottosegretaria Siracusano, il sottosegretario Freni e il ministro Fitto per la collaborazione in Commissione.

non ci siano più dubbi sul fatto che questo è il Governo delle contraddizioni. Tramite lei, signora Presidente, vorrei rivolgere l'attenzione ai colleghi di maggioranza. Siamo stati per mesi in Commissione, quando si trattava l'autonomia differenziata, a parlare di quanto tragica fosse la situazione delle Regioni italiane, di quali fossero i divari territoriali e di come ci fosse bisogno di coesione territoriale. Quando abbiamo parlato di autonomia differenziata, abbiamo spiegato quanto fossero urgenti interventi soprattutto per la perequazione infrastrutturale. Abbiamo spiegato che tante Regioni non riescono a essere attrattive proprio per le carenze infrastrutturali.

Presidente, sono rimasto un po' stupito da quello che pensavo fosse un *revirement*; pensavo che magari prima non c'erano i soldi, ma ora li hanno trovati, hanno trovato qualche soldo - anzi, 13 miliardi - per costruire un ponte, che sembra più un'opera propagandistica che una realmente e concretamente realizzabile in tempi brevi. però quei 13 miliardi li aveste distribuiti in maniera più capillare, magari avreste risolto piccole criticità territoriali. Ci sono alcune aree di crisi industriale complessa in cui con qualche milione di euro riuscireste a risolvere problemi e a creare sviluppo e occupazione.

Sembra che non abbiate ancora capito da cosa dipendono le divergenze territoriali: uno Stato che investe sempre e solo in alcune Regioni, e solo in alcune Regioni rende possibili gli investimenti, ma lascia indietro le altre, ha l'obbligo morale di pareggiare i conti; prima ancora di pensare all'autonomia, occorre fare gli stessi investimenti e far sì che ogni angolo del Paese possa avere le stesse opportunità di sviluppo.

di una politica basata solo sugli incentivi e ha creato nel tempo un disastro: mi riferisco a un'area di transizione che per anni ha beneficiato di alcuni incentivi, ed è quindi nata una zona industriale, che adesso è diventata area di crisi industriale complessa. Questa zona industriale è nata senza un progetto industriale organico, con aziende che non avevano nulla a che fare l'una con l'altra; non c'era un progetto che ipotizzava un distretto industriale. Soltanto incentivi,

le imprese sono andate via e oggi abbiamo a che fare con decine di migliaia di disoccupati per una politica che si è disinteressata di quel territorio, ma si è limitata a fare gli incentivi e poi, quando sono finiti, si è disinteressata di quell'area, che ancora oggi è di crisi industriale complessa. Se non volete ascoltare le parole che vi stiamo cercando di indirizzare, provate allora ad andare a lezione almeno dall'Europa e vedete cosa fanno gli altri Paesi. Vi abbiamo parlato

investe nelle infrastrutture. Voi su questo avete detto di no e non potete limitarvi a dare dei contentini. Dovete cominciare a pensare avendo una visione diversa sul futuro dell'Italia, se davvero avete a cuore l'intero Paese. State parlando soltanto a livello teorico, quindi utilizzando il *nomen iuris*, con il quale però posso anche vendervi un triciclo e dire che è una motocicletta, salvo poi che chi la compra si accorge che ci sono i pedali, non si va a motore e quindi non è una motocicletta. Voglio capire se vi siete resi conto delle ricadute territoriali che hanno le vostre politiche. Voi parlate agli imprenditori. Mi fa piacere che parliate agli imprenditori, ma avete capito che serve un contesto favorevole agli investimenti? Lasciamo da parte, per un momento, le infrastrutture. Avete fatto l'autonomia differenziata, quindi state navigando nella direzione opposta alla coesione territoriale. Ma voi pensate al fatto che le imprese hanno bisogno anche di un contesto di legalità? Le imprese, infatti, soprattutto gli investitori esteri, se non hanno un contesto di legalità, in Italia non vengono a investire. E voi cosa fate per creare questo contesto di legalità? Spaventate i cittadini, come se tutte le procure stessero a guardare i loro cellulari, le depotenziate, riducete la possibilità di fare delle intercettazioni. Questo è il contesto di legalità che volete creare per attirare investimenti? poi, della certezza del diritto. Anche in questo contesto tante aziende (e mi riferisco anche a quelle che se ne sono andate dal territorio in cui io vivo) vogliono certezza del diritto. Pensate alle aziende che lavorano in più ambiti territoriali. Voi qui state moltiplicando le fonti normative. Si arriverà a poter normare in maniera divergente anche fino a ventitré materie. Ma quale imprenditore deciderà di investire in Italia se deve coprire l'intero territorio nazionale? Dovrà avere a che fare con un diritto frammentario. Poi proponete la vostra stravagante soluzione di eliminare non si sa quante vecchie leggi senza neppure porvi il problema di controllare se quelle vecchie leggi ne avevano abrogate altre a loro volta. Non è questo il modo di creare la certezza del diritto. La certezza del diritto si crea se c'è un'uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Quello che state facendo ha delle ricadute territoriali pesantissime. Questo le persone, prima o poi, lo capiranno da sole e lo capiranno quando si accorgeranno che, con la cessione delle materie, tante delle risorse economiche rimarranno nelle Regioni in cui ci sono le sedi legali. Penso alle aziende che hanno la sede legale in una Regione e che lavorano in tutte le altre, magari creando ricchezza. Immagino, un'azienda che si occupa di turismo, che ha una rete di villaggi turistici nel Centro-Sud e la sede legale al Nord. Dove andranno a finire queste risorse? Dove andrà a finire il frutto di questa fiscalità? La ricchezza sarà prodotta nelle Regioni del Sud, ma andrà a andrà a finanziare le materie che vengono cedute alle Regioni del Nord. Allora, se davvero volete parlare di decreto coesione, dimostrate coerenza. Volete la coesione territoriale? Allora dovete aggiungere poco a questa norma. Aggiungete un solo articolo che abroghi l'autonomia differenziata e che spinga sulla perequazione infrastrutturale.

ringrazio il relatore, collega Gelmetti, per aver ricordato i lavori della Commissione. Egli ha affermato che i lavori si sono svolti in estrema armonia; io direi che si sono svolti nel rispetto istituzionale, anche grazie al lavoro svolto dal presidente Calandrini, ma noi, con estrema armonia, abbiamo detto di no a questo decreto-legge. Abbiamo detto di no a diversi emendamenti e confermiamo la nostra piena contrarietà a questo impianto. Quindi, si può essere armoniosi, restando risolutamente Le ragioni sono state in parte esposte dal collega che mi ha preceduto. In questa impostazione, signor Ministro, come abbiamo detto tante volte, è mancata

la provenienza, perché sono entrambe fonti di finanziamento europee, ma sono fondi che hanno anche finalità completamente diverse. Lei ha impostato il lavoro del Governo sul PNRR e sul decreto-legge

Quello che è importante a livello di coordinamento è l'idea della complementarità nelle forme di investimento (quello sì), perché quando si programmano degli investimenti, anche se si hanno fonti diverse di finanziamento, se insistono nel medesimo territorio, tali fonti debbono trovare una complementarietà

e una spinta all'accentramento. Le politiche di coesione europee nascono dall'idea molto precisa di superare i divari tra le Regioni, di arrivare ad una convergenza

o una politica di coordinamento centrale) si è sempre basato su due opposte esigenze. Quando parliamo di decentramento, facciamo riferimento ad un'idea molto particolare, cioè che le informazioni (di questo parlava già Von Hayek, lo dico ai residui liberali della destra) sono disperse nella società, quindi più noi decentriamo le decisioni e il coinvolgimento amministrativo, più siamo capaci di ascoltare i territori. D'altra parte, l'accentramento ha l'esigenza di coordinare proprio le attività decentrate e quindi tra le due opzioni ci deve essere un elemento di complementarità, da una parte, ma dall'altra anche alcuni elementi di selettività che stabiliscano le priorità. Quello che noi osserviamo da un anno a questa parte è una cascata di iniziative, fra revisione del PNRR e delle politiche di coesione, che non danno alcuna complementarità fra accentramento e decentramento, in cui c'è solo una forte spinta all'accentramento, una riduzione del coinvolgimento dei territori, ma soprattutto una forte capacità, da parte del Governo centrale, di riscrivere e determinare delle risorse che, invece, secondo la programmazione europea (mi riferisco al Fondo per lo sviluppo e la coesione) sono destinate alle Regioni e lo sono, tra l'altro, con una precisa

Cosa assume priorità? Come decide il Governo se favorire un investimento in una Regione o in un'altra? Come viene coinvolta la comunità locale? Tutte queste domande hanno ricevuto risposte

il principio, di cui abbiamo parlato tante volte anche qui in Aula col Ministro, del definanziamento, per cui alcune misure vengono spostate da una tipologia di finanziamento ad un'altra e riguardano quasi tutte il Sud.

perché in realtà il disegno del PNRR era di altro tipo: era quello di destinare - infatti la missione 1 lo faceva - tantissime risorse al potenziamento della capacità amministrativa. Dal 2008 al 2030

Il provvedimento è pieno - ne parlerà la collega Lorenzin - di misure particolari di piccole assunzioni di potenziamento del Governo centrale - qualcuno lo ha commentato come bulimia amministrativa - ma non si capisce per quale ragione il trasferimento di queste competenze di per sé dovrebbe risolvere alcuni problemi. Invece, signor Ministro, le devo dire che siamo rimasti molto delusi perché anche nella strategia emendativa

occorre individuare quali sono gli specifici svantaggi dell'insularità, non si tratta semplicemente di dire la stessa cosa in modo diverso, ma occorre definire anche a livello europeo una nuova strategia. C'è un altro tema che abbiamo posto e che invece è stato bocciato a proposito di coesione: un emendamento che destinava 800 milioni alla Sardegna e alla Sicilia per contrastare la gravissima emergenza della siccità che stiamo vivendo. In questo momento, come sapete,

siccità, circa 93 Comuni vedono interrotta la somministrazione di acqua potabile e rispetto a danni che sono stati stimati fra uno e due miliardi, abbiamo uno stanziamento di appena 20 milioni. Come mai, a proposito di coesione, non si è ritenuto necessario dire qualcosa su questo e il nostro emendamento è stato bocciato? Se la coesione e l'accentramento previsti non servono a velocizzare strade preferenziali e quindi a contrastare le emergenze che ci sono come quella della siccità in questo momento, a cosa serve questo accentramento, se non semplicemente a dare maggiori poteri e a redistribuirli anche sotto forma di consolidamento politico? Questo, signor Ministro, Ministro, è solo un esempio di come questo tipo di provvedimento sembra cadere in un momento in cui va tutto bene, in un momento di fortuna in cui ci mettiamo a ridisegnare la *governance* perché tutto il resto va talmente bene che pensiamo semplicemente a concentrarci sui meccanismi amministrativi. In realtà non è così, siamo pieni di emergenze ed effettivamente parlare di un decreto coesione nel momento stesso in cui questa maggioranza approva l'autonomia differenziata e poi risponde con un accentramento del potere, sa non soltanto di paradosso, ma in qualche modo di beffa. Ma insomma, la coesione, almeno voi della maggioranza, ce l'avete? Pensate ad uno Stato che deve avere la capacità di accentrare per realizzare delle politiche o credete nell'autonomia delle Regioni? Qui si fa tutto a stagioni alterne, in funzione del provvedimento, signor Presidente, e la cosa più triste è che noi siamo qui a rincorrere provvedimenti amministrativi di fronte ad un Paese più povero, più diviso, più bisognoso e sempre più in emergenza. Grazie Ministri, onorevoli colleghi, con il decreto che oggi ci accingiamo ad approvare si è compiuto un ulteriore passo per il rilancio delle politiche del Governo Meloni in materia di coesione economica e territoriale, un processo di riforma già avviato con l'approvazione del decreto PNRR, che aboliva l'Agenzia della coesione territoriale, e proseguito dal decreto Sud, che ha riformato il Fondo sviluppo e coesione e le ZES. Con la riforma del Fondo abbiamo introdotto lo strumento dell'Accordo per la coesione, dove le intese firmate in ciascuna Regione dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione rappresenteranno lo strumento indispensabile per sbloccare l'assegnazione alle amministrazioni regionali delle risorse. Con la riforma delle otto precedenti ripartizioni attive dal 2021, prima concentrate e legate alle infrastrutture portuali, abbiamo oggi finalmente una zona economica speciale unica che copre l'intero Mezzogiorno, con un ruolo di incentivo agli investimenti locali e di attrazione di capitali esteri. Quindi, colleghi, abbiamo un Sud non più diviso in figli e figliastri, ma con un credito d'imposta eguale per tutti, con l'importantissimo scopo di favorire volumi di investimento maggiori rispetto a quelli che le imprese meridionali avrebbero realizzato anche in sua assenza. Nella ZES il commercio e l'investimento estero giocano contemporaneamente, quindi un Governo più che avveduto ha inteso ampliare questo strumento per utilizzarlo in maniera strategica sia come vettore di interessi nazionali che per assicurare tecnologia, infrastrutture, formazione professionale a vantaggio delle società e dei territori, per farlo diventare il motore dinamico delle economie locali. La crescita del flusso delle merci e del traffico *roll on-roll off* nel Mediterraneo generato dal raddoppio del Canale di Suez rappresenterà il futuro che maggiormente andrà ad incidere sullo sviluppo del trasporto marittimo, ovviamente non appena si supererà la crisi del Medio Oriente e si tornerà alla normalità, e quindi torneremo al transito del 12 per cento di traffico mercantile mondiale e al 40 per cento di quello nazionale nazionale (un bacino di utenza enorme per le nostre aziende). Grazie al Governo Meloni, l'Italia portuale si farà trovare pronta. Il passaggio però più consistente per le politiche di coesione rimane il testo che oggi andiamo ad affrontare, il cui principio ispiratore è innanzitutto un massimo coordinamento tra gli interventi finanziati dalla politica di coesione, quelli del PNRR e della politica industriale, e dove l'obiettivo è armonizzarli tutti perché le azioni non si sovrappongano, non vadano in contrasto e non risultino conseguentemente poco efficaci. pertanto una cabina di regia per assicurare il coordinamento, salvaguardare la coerenza degli interventi finanziati, identificare le priorità delle piattaforme STEP da sostenere con il concorso della politica di coesione. In particolare, con le STEP stabiliamo che parte dei fondi da investire in questa piattaforma possano provenire da una riprogrammazione delle risorse di coesione, ossia dirottando parte di questi soldi per finanziare la politica industriale e strategica. unitarietà di sistema e una visione comune alle principali leve di sviluppo e organicità, accelerando e rafforzando l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, che aveva aveva visto finora impegni e spese quasi pari a zero. Il nostro obiettivo è invece rimettere in moto, in modo concreto, coerente e concordato con gli altri programmi, risorse europee pari a 43 miliardi di euro; a questi si aggiungono risorse di cofinanziamento nazionali e regionali per un totale complessivo di 74 miliardi. Ai soliti detrattori che non hanno saputo far altro che esprimere preoccupazione per la gestione di questi soldi rispondiamo che il decreto prevede specifiche disposizioni per garantire che ogni euro venga speso con la massima efficacia. Abbiamo messo in moto meccanismi di monitoraggio rigorosi ed incentivi per le amministrazioni regionali che rispettano i tempi e gli obiettivi previsti. Inoltre, l'introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento dimostra la nostra determinazione a non lasciare nulla al caso. Qualcuno si è detto preoccupato riguardo alla complessità burocratica e alla possibilità che le amministrazioni locali possono avere difficoltà a gestire i progetti. Su questo punto il decreto-legge in esame prevede un rafforzamento significativo della capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti; saranno organizzati corsi di formazione, supporto tecnico, ma soprattutto, con l'approvazione in Commissione bilancio del Senato dell'emendamento dei relatori, vengono stanziati 1,33 milioni per assumere 245 segretari comunali e provinciali. La modifica normativa porterà quindi a riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, ma soprattutto rappresenta un impegno concreto e tangibile per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e per consentire loro il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Ho sentito poi anche molte critiche sulla scelta dei settori strategici su cui concentrarsi. Alcuni sostengono che avremmo dovuto focalizzarci su altri. Bene, vorrei ricordare che questi settori sono stati scelti in accordo con la Commissione europea e rispondono alle necessità urgenti e alle sfide future del nostro Paese. Investire in queste aree non solo ci permetterà di rispettare le cosiddette condizioni abilitanti del regolamento europeo sulla politica di coesione, ma anche di garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti. Tutte misure, quindi, studiate attentamente per garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente e mirato, riducendo la burocrazia e favorendo una rapida attuazione dei progetti. Ma credo che la parte più bella di questo decreto si chiami Bagnoli. Per chi diceva che ci siamo fatti vedere solo a Caivano e che non ci occupiamo di tutto il resto, ecco, con questo decreto siamo arrivati anche a Bagnoli prevedendo 1,2 miliardi per la bonifica e il recupero dell'area di Bagnoli a Napoli. Questo finanziamento pertanto non ha solo una valenza ambientale, ma anche sociale, economica e di prospettiva per quel territorio e rappresenta un segnale molto significativo che mette in moto la quota dell'FSC, consentendo di arrivare a questi interventi. Con buona pace - possiamo dirlo - del presidente De Luca, che piuttosto che parlare scompostamente ogni volta che gli è possibile, dovrebbe raccontarci cosa ha fatto lui di concreto per Bagnoli *(Applausi)*, per Caivano e per il resto della Campania, visto che la governa ormai da quasi dieci anni. In conclusione, il decreto coesione rappresenta un'opportunità unica per il nostro Paese, una risposta concreta alle sfide che affrontiamo e una dimostrazione della volontà di questa maggioranza di costruire un'Italia più equa, più prospera, più unita e quindi più stabile economicamente. Vorrei da ultimo - *last but not least* - ringraziare il ministro Fitto per la pragmaticità e la concretezza messe in campo, il sottosegretario Siracusano per la disponibilità e la grande diplomazia e tutti i colleghi della Commissione bilancio per il grande lavoro svolto. Sono fiduciosa e convinta che questo decreto sia un passo nella giusta direzione e che, con grande determinazione e realismo, possiamo realizzare gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati, in nome dell'Italia tutta.

un clima civile a questo provvedimento e ringrazio per questo il presidente Calandrini e anche il ministro Fitto, con cui abbiamo avuto sicuramente una proficua interlocuzione. Questo però non toglie il fatto che i dubbi iniziali che avevamo su questo provvedimento purtroppo rimangono. Rimane non tanto la questione di fondo, il tema che sicuramente tutti vogliamo affrontare, cioè la necessità di un'armonizzazione

come opposizione, abbiamo lavorato con uno spirito totalmente costruttivo e non ostruzionistico a questo provvedimento. Però i dubbi che abbiamo avuto sin dall'inizio e che sinceramente non sono ancora venuti meno, riguardano innanzitutto il fatto che questo provvedimento tende a concludere un percorso che il Governo ha dichiaratamente già iniziato nel 2023, un percorso di accentramento a Palazzo Chigi, quindi a livello centrale, di tutte le politiche di stampo europeo, politiche che tra loro hanno origini e obiettivi molto diversificati. Sappiamo bene che i fondi di coesione mirano all'eliminazione delle diseguaglianze territoriali, tant'è vero che sono concentrati principalmente al Sud. Lo dico con buona pace della senatrice Pellegrino, perché se da Caivano si va a Bagnoli abbiamo fatto un pezzettino nella stessa Regione, ma non mi sembra una cosa eccezionale dal punto di vista delle misure di coesione. Abbiamo poi la questione che il PNRR mira ad una strategia puramente industriale e in capo ad una dimensione centralizzata fin dal suo inizio. Quindi, innanzitutto, andiamo a realizzare l'ennesima cabina di regia che si riposiziona a livello di Palazzo Chigi, con un accentramento a Palazzo Chigi e presso il Ministero di competenza di tutte le funzioni relative alle politiche del territorio, con un'azione di discrezionalità molto alta. Tant'è vero che all'inizio di questo provvedimento - e sono stati accolti, per fortuna, i nostri emendamenti - non c'erano i Comuni, non c'era la partecipazione degli enti territoriali, non c'era neanche la partecipazione, nelle fasi di azione sulle diverse competenze di questo decreto, dei soggetti di partenariato privato: pensiamo al ruolo dell'industria in tutta la parte dello sviluppo del Sud, così come delle azioni Quindi, all'inizio, la visione che ci è stata presentata dal Governo era quella di un accentramento di tutte le funzioni in questa cabina di regia, con un'azione discrezionale

che da sempre sono un elemento di criticità nella realizzazione degli interventi, rimangono depotenziate. Abbiamo ancora una questione che rimane irrisolta in questo provvedimento, che è quella del capitale umano, che è stata sollevata anche negli interventi che mi hanno preceduto, perché se

che dovranno gestire le gare e i progetti, secondo un calcolo becero che abbiamo fatto in Commissione bilancio tra quanto vengono remunerati e le risorse a disposizione, sicuramente non sono adeguati alla richiesta di competenze e di specificità che la che la complessità di questi stessi progetti richiede. Con un personale sottopagato andiamo poco lontano. Innanzitutto, non lo troviamo nella pubblica amministrazione, dopodiché non ha le qualità per portare avanti progetti coordinati da 74 miliardi. Rimane quindi una problematica

che abbiamo in campo, ma anche per immaginare processi di partenariato e di messa a terra dei bisogni strategici che abbiamo, dalle infrastrutture all'assetto idrogeologico, ai sistemi digitali,

questo provvedimento riguardava tantissimo la Commissione lavoro per il modo in cui si interviene sui contratti, su alcune aree (pensiamo a tutta la parte dell'autoimpiego, alla parte dei giovani e alla parte delle donne), in cui, a nostro parere, c'era frammentarietà degli interventi. Ancora una volta, c'era frammentarietà di interventi e non una visione che ci portasse nel medio-lungo periodo, fermo restando che Resto al Sud, che è l'altro grande provvedimento, si avvia verso la fine. Quindi, noi abbiamo una situazione dove al Sud alcuni provvedimenti che dovevano durare, soprattutto sul lavoro e sugli incentivi, fino al 2029, vedranno la fine a metà di quest'anno. Come si parlano

di impiego e di incentivo industriale nel nostro Meridione, che dovevano durare fino al 2029. Questa rimane una partita aperta, per la quale in questo provvedimento ancora non vediamo una soluzione. L'altro aspetto è quello delle cabine di regia.

però è stato un mese in Commissione, possibile che il MEF e gli altri non si parlino? Questo è un grande tema - a proposito delle cabine di regia - in cui la prima regia la dovremmo fare fra di noi, nel senso di mettere le persone intorno a un tavolo e riuscire a farle parlare. In Italia purtroppo tale questione è sempre aperta. L'altra questione che ci ha lasciato l'amaro in bocca, signora Presidente, è il fatto che non sono stati approvati i nostri emendamenti, perché chiedevamo che il Parlamento avesse una funzione. Nel momento in cui si riaccentrano le politiche a livello centrale, il Parlamento deve avere una capacità di *check and balance*, quindi la possibilità di fare un monitoraggio e che ci sia la valutazione d'impatto del monitoraggio del Parlamento almeno una volta all'anno, come abbiamo detto. *(Applausi)*. Se siete così convinti che questo nuovo modello organizzativo organizzativo porti risultati, perché non possiamo presentarlo al Parlamento? Qual è la nostra funzione? Che problema c'è a fare in modo che il Parlamento abbia contezza di come vengono spese le risorse e del cronoprogramma degli interventi attuati in una nuova strategia

Questo è un ruolo che spetta al Parlamento, a proposito di tutto il dibattito che abbiamo fatto fino alla scorsa settimana sul premierato e sul ruolo di *check and balance*. Mi avvio a concludere, però tale questione è stata non

la strada della superautonomia differenziata. *(Applausi)*. Questi due aspetti non sono conciliabili o quantomeno non abbiamo di fronte a noi un disegno unitario che ci spieghi bene cosa accadrà delle varie funzioni e dei vari livelli dello Stato e dei provvedimenti e delle azioni che mettiamo in campo nei prossimi anni con il sovraffollamento, ma anche la sovrapposizione di strumenti molto diversi fra di loro e che spesso sembrano inconciliabili.

percorso che questo Governo ha intrapreso dall'inizio della sua legislatura: un percorso che, devo dire, viene perseguito con ostinazione e soprattutto con brutale indifferenza a quelli che sono i tentativi delle opposizioni di apportare dei correttivi o quantomeno dei suggerimenti o qualcosa su cui possa valere la pena di stimolare una riflessione. Dico questo perché abbiamo già fatto presente, nell'ambito delle discussioni che hanno preceduto questo disegno di legge e hanno riguardato i provvedimenti che lo hanno preceduto, come il Governo abbia in qualche modo mutuato il sistema di controllo del PNRR che, un cosiddetto Piano per *performance*, cioè un piano di investimento dove l'erogazione delle somme è sottoposta alla verifica e al controllo del raggiungimento dell'obiettivo e, quindi, l'erogazione è scaglionata a seguito di un monitoraggio e ha deciso e ha deciso di adoperarlo anche per la gestione degli altri fondi, in questo caso il Fondo di sviluppo e coesione e anche tutti gli altri fondi di cui in questo testo si tenta di fare una sorta di armonizzazione. Ma c'è un "ma" molto grande, sul quale evidentemente non riusciamo a trovare con il Governo un punto di caduta comune che ci faccia ragionare. Nel momento Nel momento in cui si decide di mutuare lo stesso strumento di gestione del Fondo per fondi che hanno natura diversa, derivazione ed origine diversa, finalità diversa, ovviamente si comincia a creare una sorta di sovrapposizione di piani. Ma siete ovviamente consapevoli di questo nella misura in cui, con questo decreto, altro non volete fare che, appunto, cercare di dare una disciplina ed evitare l'affastellamento. Tale affastellamento, purtroppo, l'avete generato voi stessi e, soprattutto, lo ha generato il Ministro, in occasione delle varie rimodulazioni del PNRR, quando ha ha eliminato alcuni progetti dal PNRR. Mi riferisco agli interventi di rigenerazione urbana; ha promesso che comunque i progetti sarebbero stati finanziati con altre fonti; ci ha tenuti fermi otto mesi su questo argomento senza dichiarare quali sarebbero state queste fonti di finanziamento; ha sostanzialmente litigato col ministro Giorgetti, che si è rifiutato di mettere a disposizione le somme del Fondo complementare e infine, li ha reinseriti facendoli gravare prevalentemente sul Fondo di sviluppo e coesione. Siccome tutto questo non bastava a soddisfare l'azione del Governo, ha anche rafforzato i poteri di gestione centralizzata di queste fonti di finanziamento, stabilendo addirittura un superamento del potere di veto e di commissariamento degli enti locali. Cioè, se ti sta bene lo fai, come dico io, nei tempi che dico io; se non ti sta bene, ti commissario; se l'intervento è fattibile, bene, altrimenti ritiro il finanziamento queste somme le utilizzo in altro modo per altre progettualità. Come si può porre tutta questa visione, tutta quest'architrave che viene continuamente amentata e implementata con provvedimenti, circolari e DPCM? Come si può

dei lavoratori da parte delle imprese che si insediano nella ZES unica del Mezzogiorno, che possono beneficiare di uno sgravo contributivo al 100 per cento per i primi due anni, a condizione che gli assunti abbiano un'età superiore ai trentacinque

anni. Questa è una sovrapposizione di strumenti e di norme che alla fine tradisce una massificazione, una improvvisazione negli strumenti. Non c'è una strategia, non c'è una regia: c'è un tentativo semplice - per carità anche comprensibile per certi versi, ma non giustificabile - di gestire fonti di finanziamento imponenti che vengono e derivano da finalità diverse, che il Governo ha invece tirato tutte insieme all'interno di un unico calderone e che adesso deve incominciare a dipanare. Si è, infatti, creata una grandissima confusione:

con amarezza perché abbiamo denunciato nella legge di bilancio che il fondo perequativo, cioè il fondo destinato al Sud, era stato svuotato e vi erano rimasti appena 800 milioni. Tuttavia, su questo rilievo io rammento il silenzio assoluto da parte tanto del Governo e delle forze della maggioranza.

con la piena conferma che fino adesso era stato sostanzialmente svuotato a favore di altri interventi, fatti in altri posti, sicuramente non nel Sud Italia. Non ci consola neppure che sia stato previsto uno stanziamento *standard* del 40 per cento delle risorse a valere sui fondi di bilancio per gli interventi al Sud, perché questa non è

e non mantenendo i vincoli sui fondi per lo sviluppo e la coesione: perché questi ultimi sono maggiori di quelli di bilancio, perché questi ultimi sono più vincolanti e gli altri li possiamo cambiare?

ma assolutamente non puntuale, purtroppo. Anche su questi interventi ci aspettiamo una risposta, ma purtroppo sappiamo già che tarderà ad arrivare o addirittura mancherà del tutto. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni.

che promette dal titolo di risolvere una serie di questioni e poi si smentisce sostanzialmente nei contenuti. In questo decreto-legge ci sono molte cose che non ci piacciono, ma sulla prima, che è la più importante, vorrei spendere qualche minuto. Si tratta di un decreto-legge che affronta in modo del tutto inadeguato la questione fondamentale della coesione nel nostro Paese. Una settimana fa, la Commissione europea ha rivolto un monito al nostro Paese perché acceleri la discussione sull'attuazione dei programmi di politica di coesione sociale insieme al rafforzamento delle capacità amministrative a livello nazionale, in particolare a livello subnazionale. La Commissione europea ha sottolineato delle cose che sostanzialmente il ritardo economico del Mezzogiorno rappresenta la più importante fonte di disuguaglianza per l'Italia e uno dei maggiori freni per la crescita economica complessiva del Paese.

Basti vedere la spesa pubblica *pro capite*: nel Nord-Est si registra una spesa più alta, 197 euro *pro capite*, quasi tre volte superiore a quella del Sud, che è di 72 euro. La spesa dei Comuni della Calabria, ad esempio, è di 37 euro *pro capite*

in particolare tra Nord e Sud del Paese, ma questo lo si è visto anche con i finanziamenti del PNRR; in Italia abbiamo avuto più finanziamenti perché era necessario affrontare il problema delle disuguaglianze nel Paese.

dei fatti, occorrono degli interventi normativi. Invece assistiamo sostanzialmente a dei *bonus*, ad assunzioni precarie: cioè non c'è un'idea

e si va avanti così, ma questo non crea coesione sociale. Nello stesso tempo, in Parlamento sono state approvate - lo hanno già detto altri - politiche

Già altri hanno ricordato che, se abbiamo recuperato nella *governance* la partecipazione dei Comuni e delle autonomie locali, è stato solo grazie ad emendamenti che abbiamo presentato. Avete però lasciato fuori le parti sociali, che sono fondamentali almeno a mio avviso - per affrontare il problema della questione sia del governo dei processi di trasformazione, sia degli indirizzi di politica industriale, economica e turistica.

il dato che non ci convince ed è per questo che diamo un giudizio negativo sia sul merito che sul metodo. La questione

intervengo con piacere oggi sul decreto-legge coesione che riguarda il Mezzogiorno, il lavoro dei giovani e delle donne e affronta numerose altre questioni legate all'utilizzo più puntuale dei fondi europei e nazionali per la coesione territoriale. Mi stimola anche l'intervento del collega Magni, che ha parlato del concetto di coesione e lo ha messo in contrapposizione all'autonomia differenziata alla situazione che c'è nel Mezzogiorno. In realtà è vero: la parola coesione è bella; deriva dal latino *coesus* e significa stare insieme, essere uniti. Richiama alla mente immagini di unione, di armonia, di concordia e il desiderio umano di integrazione, dove gli elementi si legano tra di loro per creare un'unità più forte e stabile. In fisica la coesione descrive la forza che tiene insieme le molecole di un materiale, determinandone la resistenza e la stabilità. Ad esempio, la coesione dell'acqua permette alle gocce di formarsi e muoversi verso l'alto di un tubo, superando la forza di gravità. Allo stesso modo, la coesione tra le persone in una comunità permette loro di sostenersi a vicenda, di aderire a valori condivisi e di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, superando gli ostacoli, proprio come le molecole d'acqua. Quindi, la coesione non è solo un principio economico, non può riguardare solo gli aspetti economici, ma è un valore culturale e politico, che ha radici profonde e ha un senso di identità nella nostra storia. rappresenta un elemento fondamentale, riferito proprio al Mezzogiorno, per rafforzare il tessuto sociale ed economico del Paese, soprattutto delle Regioni più svantaggiate. Significa solidarietà, che è necessaria per superare le disparità, e permette a una nazione di affrontare sfide globali, con una visione condivisa del futuro. In questo decreto-legge ci sono misure importanti, che sono state sottolineate prima dai colleghi. Ci sono contributi per gli *under* 35 e sgravi fiscali; c'è Resto al Sud, con contributi a fondo perduto per promuovere nuove attività imprenditoriali, specialmente nel Sud.

provvedimento e riguardano l'impiego delle risorse in settori più strategici, come le infrastrutture per il rischio idrogeologico, la protezione dell'ambiente, le risorse idriche, i rifiuti, i trasporti, la mobilità sostenibile, l'energia, la transizione digitale e la transizione verde, il sostegno alle attività di impresa. Si tratta di una serie di programmi di investimento per complessivi 74 miliardi di euro, finanziati con risorse europee,

la coesione del nostro Paese con il voto dato qui in Senato sulla legge sull'autonomia differenziata. Siamo stati accusati, con tanto di manifesti pubblicati e affissi sui muri e sui cassonetti stradali delle nostre città, città, di tradimento del nostro territorio e di aver voltato le spalle al Sud. Eppure, qui in Senato abbiamo lavorato intensamente per modificare il testo originario di quella legge presentata dal ministro Calderoli, inserendo norme specifiche che tutelano il Sud. Con le modifiche introdotte, nessuna delega di autonomia potrà essere attuata senza prima garantire la definizione, la quantificazione e soprattutto il finanziamento dei LEP, che sono riferiti ai diritti sociali di tutti gli italiani, e quelli civili credo siano già garantiti. Le accuse a noi rivolte sono state alimentate da quelle forze politiche, cui si sono uniti anche dei vescovi del nostro territorio, che nel 2001 promossero la riforma del Titolo V, consentendo alle Regioni di gestire la quasi totalità dei servizi, senza garanzie di rispetto, senza l'accenno a una benché minima idea di livello minimo essenziale e senza riferimento alcuno ai LEP. Oggi, grazie alla legge sull'autonomia, il nostro impegno può essere la garanzia che il Sud dell'Italia potrà fare un passo avanti. il meccanismo che abbiamo introdotto garantisce una distribuzione più equa a patto che i LEP siano adeguatamente finanziati. Questa sarà la vera rivoluzione culturale del nostro Paese: bilanciare i servizi essenziali, oggi carenti in alcune aree, specialmente al Sud, rappresenta un'opportunità per unire l'Italia attraverso l'equità. Questa è la vera coesione e dice il giusto chi sostiene che non c'è necessità di accelerare questo processo di approvazione definitiva, anche del testo di quella legge alla Camera, dato che oggi non si vede all'orizzonte la possibilità di finanziamento dei LEP. E, senza il finanziamento, quella legge rimarrà sostanzialmente inapplicabile, diventando un argomento divisivo per il nostro Paese, che nella sostanza è stato sempre diviso e c'è sempre stata la questione meridionale: un Paese diviso fra Nord e Sud. Per lo stesso motivo dico che ha ragione il nostro segretario Tajani quando dice che è necessaria una vigilanza attiva sull'applicazione di quella legge, garantendo ogni nuova iniziativa che possa essere di autonomia data alle Regioni solo dopo aver messo sullo stesso piano i territori, con una partenza uguale per tutti con riguardo ai servizi essenziali che interessano tutti i cittadini. Ci vuole la vigilanza attiva: abbiamo visto altre leggi nel passato, tantissime, che sono partite con l'obiettivo di creare sviluppo al Sud e hanno prodotto risultati opposti. Ricordo per esempio la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che ha lasciato un elenco interminabile - alcune situazioni vengono riprese proprio con questo decreto coesione coesione - di fallimenti industriali legati a una cattiva visione strategica, con bonifiche poi da effettuare sul territorio. Penso all'industria petrolchimica di Manfredonia, all'industria siderurgica di Gioia Tauro, quella chimica di Saline Joniche, alla Liquichimica di Salerno, allo zuccherificio di Termoli, alla Liquichimica di Crotone, o all'Italsider, che è trattata nel provvedimento di Bagnoli, allo zuccherificio di Policoro, all'industria del cemento di Porto Torres in Sardegna e all'industria chimica di Gela Sono esempi che riflettono problematiche comuni che hanno avuto visioni sbagliate, pur partendo da provvedimenti che avevano come interesse il il superamento del *gap* industriale, anzi economico-sociale fra Nord e Sud. Noi di Forza Italia abbiamo sempre sostenuto valori liberali, esaltando la sussidiarietà e la libertà individuale contro l'eccessivo intervento dello Stato. Ecco perché siamo per la coesione, siamo per l'etoeconomia. La nostra visione punta a un equilibrio tra l'autonomia delle Regioni e un'unità d'Italia forte e coesa. Non possiamo però ignorare che ogni decisione riguardante l'autonomia debba anche considerare l'intero tessuto nazionale. Attualmente si dice che manchino le risorse; infatti, hanno previsto per i LEP 170 miliardi di euro. Sono tanti. Ma, se pensiamo che negli ultimi anni abbiamo utilizzato per i *bonus* 150 miliardi (sono rimasti a carico degli italiani e a carico dello Stato) e 40 miliardi per il reddito di cittadinanza, capiamo che anche in prospettiva questi provvedimenti possono essere un aiuto per capire in che direzione possa andare il nostro Paese. Ovviamente sono provvedimenti che vanno supportati con risorse. Ecco perché i 170 miliardi previsti, che possono essere anche graduali, in qualche modo porterebbero all'attuazione piena di questo provvedimento e anche di quelli collegati che riguardano ovviamente il decreto di cui parliamo. Allora la nostra visione deve essere rivolta al futuro la mia esperienza di sindaco mi dice che il problema principale del Sud è la mancanza di opportunità di lavoro dei giovani. Bisogna insistere sul progetto di coesione e non ci saranno mai risorse. Forse è su queste cose che dovrebbe

è stato assegnato al Sud, che avrà anche circa l'80 per cento dei 32 miliardi assegnati alle Regioni dal Fondo di sviluppo e coesione e i 75 miliardi di euro della programmazione europea per la coesione, di cui l'85 per cento è destinato al Sud. Sud. Riusciremo a spenderli? È su questo tema che dovremmo confrontarci. Per quanto ci riguarda, il nostro impegno deve essere quello di guardare oltre le critiche immediate e lavorare per il bene comune, con la consapevolezza che le decisioni difficili di oggi saranno di oggi saranno anche i pilastri per il benessere del domani. La coesione, in fin dei conti, è l'essenza della nostra unità nazionale, è il fondamento su cui costruire un futuro per tutti noi.

poc'anzi, quando ha iniziato a parlare in discussione generale su questo decreto, ha parlato di contraddizione. E allora sul percorso delle contraddizioni che contraddistinguono questo decreto-legge proviamo a continuare e, quindi, a chiarire meglio i concetti che a noi in realtà non sono piaciuti e che però non piaceranno nemmeno agli italiani.

era prevista al 30 luglio; sapevamo perfettamente che il ministro Fitto ne voleva l'eliminazione e non voleva assolutamente che fosse prorogata; poi improvvisamente oggi leggiamo sui giornali che il Governo fa marcia indietro su quella misura che ha contribuito nel tempo

Oggi come atto dovuto leggo dai giornali che il ministro Fitto dice, contento, che per fortuna abbiamo avuto una proroga di sei mesi, ma era un atto dovuto; vedo anche un'autocelebrazione per questo motivo, ed è sui giornali.

la sede legale di chi fa impresa al Sud, prendendo gli incentivi, può essere al Nord e basta che la sede operativa sia al Sud; anche lì abbiamo quindi alcune contraddizioni abbastanza evidenti.

in altri termini, interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (nel dettaglio, nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio). Il ministro Fitto ha ribadito più volte che l'obiettivo prefissato in questo articolato è restituire ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado alle porte di Napoli e valorizzarne la posizione strategica, anche in prospettiva di un rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno, a riprova del fatto che il Governo può agire concretamente. Lo stesso Ministro poi considera il finanziamento rilevantissimo, con valenza non solo ambientale, ma anche e soprattutto sociale, economica e di prospettiva per il territorio interessato: è un segnale importante, che mette in moto la quota del Fondo sviluppo e coesione assegnata a quel territorio, che consentirà in sinergia con tutti i componenti della cabina di regia, a partire dal sindaco di Napoli, che è commissario di Bagnoli - di avviare questi interventi. Signora Presidente, se per il ministro Fitto la somma destinata a Bagnoli rappresenta un finanziamento di un certo rilievo, per noi rappresenta invece una grave mancanza, anzi gravissima, costituisce l'ennesima vergogna ammazza Sud, nient'altro che la continuazione di un'operazione scellerata di sventramento delle casse meridionali. Non può e non deve sfuggire che l'assegnazione delle risorse prevede l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione già destinati per legge alla Regione Campania: doveroso allora risulta chiederci e chiedere, se il sito è d'interesse nazionale (SIN), perché Bagnoli è un SIN, e allora perché si intende riqualificare l'area con il Fondo per lo sviluppo e la coesione e non aggiungere in realtà i fondi nazionali? Bagnoli infatti ha bisogno di altro: altro: è contigua alla zona rossa di Pozzuoli per l'area sismica e, quindi, avrà necessità di altre opere. Così abbiamo provato a inserirla all'interno degli emendamenti, in una proposta emendativa che non è passata. Bagnoli è un'area divisa da binari delle Ferrovie dello Stato e della metropolitana. In caso di bradisismo, i cittadini hanno difficoltà addirittura a raggiungere l'interno con l'area della costa. Quindi, si poteva intervenire in tal senso con i fondi di coesione. Invece no: essi vengono destinati per altre opere già previste.

Prendiamo il caso dell'ospedale di Ischia, che in settimana ha visto cedere un motore del condizionatore per le gravi inefficienze e le carenze strutturali che esso riporta, così come tanti altri ospedali. Signor Presidente, concludo ribadendo ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, che la nostra azione, come MoVimento 5 Stelle, sarà quella di monitorare affinché si smetta con violenze e scippi al Sud, soprattutto con i fondi di coesione. Basta con questo scippo! *(Applausi)*. Signora Presidente, questo provvedimento è molto articolato e affronta una pluralità di argomenti. Mi concentro su alcuni punti qualificanti, tentando di integrare le riflessioni che hanno già svolto i colleghi e le colleghe intervenuti prima di me. Il primo punto è il tema dell'accentramento delle politiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Come hanno detto altri colleghi, con questo provvedimento il Governo prosegue un'opera di accentramento dei poteri delle politiche a Palazzo Chigi che è stata messa sistematicamente in campo nei diciannove mesi di operatività del Governo Meloni. In questo caso, la centralizzazione riguarda la programmazione e l'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione. Come dicevo, è parte di un processo. Se mettiamo in fila quello che è accaduto e sta accadendo, questo dato politico diventa evidente. Pensiamo alla proliferazione delle cabine di regia, alla nascita di diversi dipartimenti. Pensiamo anche alla centralizzazione interministeriale, alla sottrazione al MEF della gestione del PNRR, che è stato portato interamente a Palazzo Chigi. Pensiamo anche a quello che sta venendo avanti, macroscopico: è il provvedimento di riforma costituzionale che introduce il premierato, con il suo carico di accentramento dei poteri nella figura del o della Presidente del Consiglio. È una tendenza solo apparentemente in contraddizione con la legge sull'autonomia differenziata, che dovrebbe portare all'attribuzione di forme ulteriori di autonomia alle Regioni che ne fanno richiesta. Parlo di apparente contraddizione, perché, in realtà, il disegno politico del Governo emerge chiaramente: l'autonomia differenziata per le Regioni ricche del Nord, che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale; la più spietata centralizzazione nei confronti delle Regioni del Mezzogiorno, con la centralizzazione della gestione della programmazione delle risorse europee nazionali; lo smantellamento delle otto zone economiche speciali centralizzate, unificate ancora una volta in capo allo Stato centrale, sulla base di un pregiudizio implicito nei confronti della classe dirigente del Mezzogiorno, che, di fatto, viene spogliata di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo; pregiudizio negativo nei confronti degli amministratori locali e degli amministratori regionali e la centralizzazione di tutte queste politiche in nome, questo sì, di un modello istituzionale differenziato e - mi sia consentito dirlo - discriminatorio. L'articolato di questo decreto-legge stabilisce che, anche per le politiche di coesione, il percorso è appunto quello dell'accentramento delle competenze e degli ambiti dei poteri decisionali nel Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le conseguenze sono lo svuotamento, il mancato coinvolgimento, l'espunzione vera e propria delle Regioni e degli enti locali dal sistema di Governo e il rifiuto, il rigetto nei confronti di qualunque ipotesi di monitoraggio parlamentare. Il ruolo che il decreto-legge in esame affida alla cabina di regia e i poteri affidati al dipartimento di fatto abbattono e ridimensionano i principi di partecipazione, di multilateralità e la *governance* multilivello, che era l'essenza delle politiche di coesione, per come sono state introdotte e implementate nel Paese. È emblematica, da questo punto di vista, la formulazione iniziale dell'articolo 3 sulla cabina di regia, dove di fatto non era previsto alcun coinvolgimento nemmeno degli enti locali; solo grazie a un nostro emendamento e alla battaglia che abbiamo condotto nella Commissione parlamentare di riferimento, il Governo

hanno funzioni ancillari rispetto alla cabina di regia, così come disegnata dal provvedimento. Il secondo punto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa, che è cruciale se vogliamo raggiungere un obiettivo condiviso, cioè un'accelerazione della spesa delle risorse europee e nazionali a disposizione per le politiche di coesione e di sviluppo. Il rafforzamento della capacità amministrativa si traduce in misure e in scelte del tutto insufficienti, come hanno sottolineato altri colleghi. Invece di proporre concorsi pubblici, che dovrebbe essere la via maestra il reclutamento nella pubblica amministrazione di quelle competenze, di quelle alte professionalità che servono per quel salto di qualità che, a parole, viene invocato come una delle ragioni fondative di questo provvedimento, la scelta è quella di assunzioni di carattere precario, di basso livello professionale e retributivo - lo ripeto - quando invece sarebbe necessaria un'operazione radicalmente diversa. Per non parlare del pannicello caldo dell'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali. Sempre in questo contesto, che noi riteniamo molto discutibile, è paradigmatica ancora una volta la scelta che si fa con la convenzione con la società *in house* Eutalia Srl, dove il reclutamento viene addirittura fatto con la compilazione di un modello e un colloquio conoscitivo; però, in caso di assenza di candidature o di candidature ritenute idonee, o di impossibilità ad assumere l'incarico da parte di soggetti ritenuti idonei, la società può comunque individuare collaboratori tramite selezione diretta. Addio a qualunque forma pubblica di reclutamento, per non parlare delle procedure concorsuali, e vai con il reclutamento diretto, evidentemente su basi assolutamente discrezionali. Avviandomi alla punto riguarda il tema del Mezzogiorno, che naturalmente è cruciale in un decreto-legge dedicato alla coesione. È stata appena approvata la legge sull'autonomia differenziata, che produrrà le conseguenze che abbiamo denunciato in quest'Aula così come alla Camera dei deputati e nel dibattito pubblico nel Paese. Questo provvedimento prosegue in un percorso di vero e proprio abbandono del Mezzogiorno d'Italia Dico ciò pensando alle disposizioni sull'assegnazione delle risorse della programmazione della politica di coesione, a quello che viene fatto sul tema delle anticipazioni. Ma penso anche alla clausola, apparentemente migliorativa, che eleva dal 34 al 40 per cento la quota di investimenti da destinare alle Regioni del Mezzogiorno; aumento, però, avviene su un perimetro ridotto rispetto a quello iniziale, perché si escludono gli investimenti di RFI e quelli di ANAS e quindi, di fatto, ci si limita agli investimenti delle amministrazioni centrali;

migliorato, dei meccanismi di monitoraggio in corso e di verifica *ex post* dell'effettivo rispetto della clausola che quantifica in questo caso nel 40 per cento la quota di investimenti da destinare al Mezzogiorno. *Dulcis in fundo* mi rivolgo al signor Ministro - veniamo alla parodia, perché questo è l'unico termine che si può utilizzare, del Fondo perequativo infrastrutturale, che è stato introdotto negli anni passati come parte attuativa della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Peccato che questo Fondo avesse 4,6 miliardi di dotazione nella versione iniziale e ne siano rimasti 700, ovvero 100 milioni all'anno dal 2027 al 2033. Si può anche ridenominarlo «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» destinando il 100 per cento di queste risorse e non l'80, come nella versione precedente, al Mezzogiorno, per cento di 700 milioni è comunque enormemente di meno dell'80 per cento di 4,6 miliardi e questo noi lo denunciamo con forza in questa sede. *(Applausi)* Vorrei proseguire, ma temo di aver esaurito il tempo, sulle disposizioni per l'autoimpiego, per le agevolazioni alle assunzioni: qui non c'è molto di nuovo rispetto al passato, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista delle risorse stanziate, anche queste misure, che sono deludenti rispetto alle aspettative e a quello che sarebbe necessario mettere in campo, confermano la valutazione negativa su questo provvedimento, su misure specifiche che contiene, ma soprattutto sulla filosofia complessiva che lo ispira.

di assenza di logica strategica, di contraddizione rispetto a un provvedimento legato alla coesione con l'approvazione dell'autonomia differenziata, tutte cose - per carità - rispettabili in quanto opinioni, ma se si vuole essere oggettivi, leggendo il provvedimento, prendere atto del lavoro che è stato svolto in Commissione, di cui hanno parlato i relatori, in cui con spirito - ritengo - assolutamente attento sono stati accolti diversi emendamenti dell'opposizione, a dimostrazione che il lavoro non è stato fatto con pregiudizialità, ma con la volontà di costruire un provvedimento veramente ben fatto e, laddove qualcuno ha fatto notare che magari c'era qualcosa da migliorare, lo si è

finalmente una politica di coesione che mette a sistema tutte le risorse disponibili che - ricordo a me stesso - sono risorse di per sé straordinarie, che quindi necessitano di un approccio straordinario e che hanno bisogno di una visione strategica per cui si fanno le cabine di regia, per cui è necessario che il potere centrale interloquisca con i vari livelli di potere locale, mantenendo la strategia. Per questo abbiamo stretto gli accordi di sviluppo e coesione: per avere un diverso rapporto con le istituzioni delle Regioni nel quale, insieme a loro, si è costruito un elenco di priorità

Grazie a tutti.

Queste sono, in estrema sintesi, le linee guida del provvedimento in esame, che intende realizzare una vera e propria riforma della politica di coesione inserita nel processo di revisione del PNRR, ciò al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 finalizzati in una nuova struttura a ridurre divari e dislivelli territoriali. Per un quadro d'insieme e una valutazione completa il decreto va quindi letto ad ampio spettro e in combinato disposto con i dettati e le riforme del PNRR, che prevede un robusto impegno normativo teso ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea. Il nuovo provvedimento, pertanto, alla luce di queste considerazioni, intende attuare le riforme previste nel PNRR muovendosi nella cornice tracciata dal decreto-legge Sud e in particolare si muove su tre indirizzi principali: le misure per attuare la riforma della politica di coesione, gli interventi per lo sviluppo, gli interventi per il lavoro. Con riferimento alla riforma della politica di coesione, il nuovo testo introduce misure per potenziare l'efficienza della spesa e aumentare la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibili. Inoltre, si intende giungere a un quadro complessivo in cui tutte le risorse del Fondo di coesione e del PNRR vengano utilizzate in maniera sinergica, al fine anche di velocizzare la procedura e migliorarne la stessa attuazione. Il sostegno allo sviluppo competitivo del sistema produttivo, soprattutto nel Mezzogiorno, è trasversale a più misure e concerne diversi fronti. Cito la dotazione infrastrutturale, con la revisione della disciplina del Fondo perequativo, specificatamente dedicato al Sud, che non era una dimenticanza: si è attesa la rivisitazione di tutte le risorse disponibili per poter avere finalmente un Fondo perequativo degno di questo nome che sicuramente attenziona i *gap* infrastrutturali nel Mezzogiorno. Quindi c'è un potenziamento dell'attività di ricerca e di innovazione, come il recupero dei siti industriali del Sud nei Comuni superiori a 5.000 abitanti. Il tema del lavoro rappresenta, negli obiettivi del Governo, l'altro capitolo portante del provvedimento in esame. In particolare, il decreto-legge introduce una serie di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, indirizzate a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti quali i giovani, le donne e i disoccupati di lunga durata. A disposizione per la promozione dell'occupazione sono previsti oltre 2,8 miliardi a valere sul programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e sulle risorse del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori. si aggiungono le risorse per la riconversione delle competenze dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi. Le misure intervengono lungo tre direttrici fondamentali. Per l'occupazione, si introducono disposizioni per incentivare l'avvio di progetti di autoimprenditorialità nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, per sostenere l'occupazione nelle ZES e favorire l'assunzione di giovani e donne; le politiche attive a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; la prevenzione e il contrasto al lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati. Al fine di incentivare nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero professionale al Centro-Nord e nel Mezzogiorno sono previste due misure specifiche dominate Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0. Beneficiati dalle stesse sono i giovani *under* 35 in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi o disoccupati, o ancora disoccupati e destinatari delle misure di politica attiva (Garanzia Sono previsti altresì finanziamenti per i servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare, di tutoraggio per l'incremento delle competenze, o veri e propri sostegni all'investimento attraverso *voucher* e interventi in regime di *de minimis*. Poi ci sono gli sgravi legati al *bonus* giovani, al *bonus* donne e tante altre misure legate sempre alle politiche attive del lavoro. La politica di questo Governo non mira al sussidio che mantiene le persone, soprattutto i giovani, in condizioni di perenne subordinazione rispetto al potere politico, ma alla dignità del lavoro che si acquisisce con gli incentivi. *(Applausi)*. Quando si parla di incentivi, non si parla di sussidi a pioggia, ma della capacità di innescare processi virtuosi che oggettivamente creino possibilità di sviluppo a lungo termine; per cui si chiamano incentivi e non sussidi. Tali interventi sul lavoro stimolano la riflessione sulla misura decontribuzione Sud, al centro del dibattito pubblico nelle scorse settimane e oggetto, come spesso accade, di imprecisioni e polemiche strumentali. È notizia odierna che, grazie al ministro Fitto, che ringraziamo, è stata ottenuta la proroga di questa importante misura al 31 dicembre di quest'anno, con una apertura da parte delle istituzioni europee sulla possibilità di renderla misura strutturale, a dimostrazione di quanto la polemica strumentale catastrofista delle opposizioni sia fallace. Non è stato certamente il Governo Meloni che voleva interromperne il rinnovo. Infatti ci siamo attivati per negoziare, sempre attraverso il ministro Fitto, con la Commissione europea nuove modalità possibili di applicazione della misura, in conformità con la disciplina europea. La misura decontribuzione Sud è stata infatti decisa dall'Europa come strumento straordinario per affrontare prima la crisi dovuta alla pandemia, poi quella correlata alla guerra in Ucraina. Non a caso, anche i Governi che ci hanno preceduto hanno potuto procedere solo attraverso proroghe di sei o di dodici mesi, proprio come il Governo Meloni. L'Europa adesso ha deciso che misure del genere debbono essere interrotte in tutti gli Stati, quindi il ministro Fitto sta tenendo aperto il dialogo con la Commissione per ottenere un'apertura un'apertura per misure analoghe, che abbiano però una natura strutturale di incentivo per i giovani, al fine di costruirsi un futuro dignitoso, e non l'ennesimo sussidio di Stato. misure in buona parte sono già previste, appunto, nel decreto coesione. Sul piano delle infrastrutture, poi, è previsto che almeno il 40 per cento delle risorse venga riservato al Sud. Non mancano gli interventi per scuole e istituti tecnici, oltre a quelli per la legalità, con i quali, ad esempio, si punta alla reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tutti interventi che rientrano nel quadro della revisione del PNRR, portata avanti con autorevolezza dal nostro Governo in Europa e in sintonia con altri provvedimenti, come la ZES unica per il Sud, una vera e propria rivoluzione che consentirà finalmente al Mezzogiorno di crescere e di colmare il divario con il resto dell'Italia e dell'Europa. L'importante lavoro svolto dal Governo Meloni, e in particolare dal ministro Fitto, è stato riconosciuto anche dalla Conferenza unificata delle Regioni e delle Province, che si è espressa favorevolmente al provvedimento. Non si tratta di un via libera di *routine*, né peraltro scontato. Il parere della Conferenza unificata segna un'ulteriore accelerazione del percorso di riforma della politica di coesione portato davanti dal ministro Fitto e dal Governo. La linea tracciata dal decreto Sud prima e dal decreto-legge coesione dopo spiega in modo assai concreto il senso del nuovo corso italiano nel campo della politica di coesione, sulla quale Bruxelles - come già detto - ha ampiamente concordato,

è stato designare una possibilità di sviluppo concreto per il nostro Paese, oggettivamente legata a una visione che altri hanno ignorato per anni, perché hanno preferito, loro sì, vivere alla giornata, vivere sul singolo intervento, vivere sulla singola elemosina concessa al Sud e soprattutto ai giovani del Sud.

Grazie, Presidente. Ho ascoltato con molta attenzione i contenuti dei vari interventi e penso che sia molto importante, in questa replica, fare due considerazioni, una di carattere generale, anche per respingere alcune critiche che sinceramente mi sembrano abbastanza ingenerose sulle scelte che il Governo ha messo in campo, e una per rispondere in modo molto puntuale e dettagliato ad alcune valutazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti. Sulla prima parte, penso che ci sia la necessità di mettere in campo qualche riflessione più specifica. Non ho ascoltato nessuna valutazione su cosa è accaduto in questi anni, non ho ascoltato nessuna valutazione e nessun giudizio sull'efficacia o meno delle politiche di coesione, cioè delle risorse europee, non ho ascoltato nessuna valutazione su quelli che sono non i giudizi della maggioranza, ma i risultati che emergono dai rapporti che la Commissione europea ha presentato, sia lo scorso anno che quest'anno. Quei rapporti indicano l'Italia come il Paese che è chiuso in una trappola di sviluppo, come il Paese che usa male le risorse che gli vengono assegnate, come il Paese che non è riuscito a rendere efficace questa spesa. Non lo diciamo noi; basta leggere questi rapporti, per capire che l'approccio sull'uso di queste risorse dovrebbe essere leggermente differente da parte del nostro Paese, essendo l'Italia uno dei principali beneficiari della politica di coesione. Lo dico anche con un altro elemento, che mi sembra molto assente dal dibattito che abbiamo tenuto, soprattutto sul fronte critico. Non ho ascoltato nessuna valutazione, ascoltato nessuna valutazione, in termini di comparazione con gli altri Paesi europei, sui rischi che corre l'Italia. Siccome siamo in una fase nella quale il prossimo bilancio europeo punterà anche all'allargamento dell'Unione europea, la politica di coesione, insieme a quella dell'agricoltura, saranno i due due capitoli del bilancio europeo più grossi e più a rischio. I Paesi come il nostro, che hanno una maggiore possibilità di utilizzo, dovrebbero essere più preoccupati della qualità della spesa. Concludo la premessa respingendo

proprio per avere una visione strategica ed evitare la sovrapposizione degli interventi e per evitare che la mano destra non sapesse quello che faceva la mano sinistra. L'abbiamo fatto anche secondo una logica che - consentitemi - ha anticipato di circa un anno le raccomandazioni della Commissione europea, che nello scorso luglio ha indicato agli Stati membri di creare una sinergia tra il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la politica di coesione. Alcuni colleghi di maggioranza - che ringrazio - hanno ripercorso le scelte che il Governo ha messo in campo: da un lato, la riforma del Fondo di sviluppo e coesione, dall'altra la revisione - per fortuna del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della sua *governance*. Dall'altro ancora, si completa con questo decreto la riforma della politica di coesione, che non è per caso, nella revisione del PNRR, una delle sette nuove riforme che abbiamo inserito, che dà proprio il "la" alla visione organica dell'utilizzo di queste risorse e mette in campo una strategia che indica in modo coordinato l'uso delle stesse risorse. Ho ascoltato un'altra critica sull'accentramento. Sinceramente la trovo paradossale, perché dei tre fondi dei quali parliamo non c'è stato alcun accentramento nel merito. nel merito. Poi, nella narrazione possiamo anche dire questo, ma quando abbiamo deciso la riforma del Fondo di sviluppo e coesione, cioè delle risorse nazionali, non abbiamo accentrato; abbiamo lasciato le risorse alle Regioni e abbiamo invertito un meccanismo, che era quello dell'assegnazione delle risorse al buio senza termini, senza progetti, senza cronoprogramma. Abbiamo obbligato a proporre delle soluzioni affiancate da un cronoprogramma temporale e finanziario per realizzare gli interventi, sottoscrivendo un'intesa. Abbiamo fatto lo stesso nell'ambito della nuova *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove non c'è un accentramento di poteri, ma c'è una organizzazione identica a quella che la Commissione europea ha messo in campo per tutti i piani nazionali di ripresa e resilienza, perché abbiamo messo di fronte allo specchio l'organizzazione europea. Abbiamo messo in campo una struttura centrale che si raccorda con le altre amministrazioni. Anche qui, devo dire, ho ascoltato critiche che non corrispondono ai contenuti del testo. Non c'è una cabina di regia che fa nuove assunzioni, com'è stato detto; c'è una cabina di regia che c'era, che utilizzava le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, che era finalizzata a quello, che si allarga alle amministrazioni interessate alla politica di coesione, cioè programmi europei di competenza nazionale, e che coinvolge al suo interno, su richiesta avanzata dopo il confronto che abbiamo avuto con l'ANCI e l'UPI, anche i loro rappresentanti, in una visione che non aggiunge nulla dal punto di vista organizzativo e che mette in campo una scelta totalmente condivisa - lo ricordava il senatore Russo poco fa -, tant'è che sinceramente è singolare ascoltare questa critica dopo un parere favorevole da parte della Conferenza unificata. Quindi, si è più realisti del re in quest'Aula, perché, anziché anziché prendere atto del fatto che, nel confronto con Regioni, Province e Comuni, si è costruita positivamente una dimensione ed una condivisione di questo testo, si indica una criticità proprio in questo pseudo-accentramento che semplicemente non esiste. Abbiamo fatto di più con questo decreto: abbiamo anche individuato delle modifiche sostanziali a programmi che sono di competenza nazionale. Per quanto riguarda i programmi regionali, vorrei capire dov'è scritto in questo decreto che il Governo accentra e toglie poteri, competenze e risorse alle Regioni. È vero il contrario. È vero che le Regioni, per poter attivare il programma di coesione di loro competenza, hanno bisogno di mettere come quota di cofinanziamento risorse che non avevano e che il Governo, prima col decreto sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per una parte, e poi con questo decreto per il suo completamento, mette a loro disposizione per poter cofinanziare questo programma, che diversamente non sarebbe partito.

che ritengo fondamentale per migliorare la qualità della spesa: le risorse per poter cofinanziare questi programmi vengono assegnate sulla base dei dei risultati raggiunti. E non è vero che non ci sono gli obiettivi, perché nei programmi regionali non imponiamo nulla: noi indichiamo le cinque priorità che sono le condizioni abilitanti indicate dalla Commissione europea nella politica di coesione, che inseriamo all'interno di questo decreto-legge e che dicono sostanzialmente che bisogna

interventi per il ciclo integrato dei rifiuti? È normale che, dal punto di vista della risorsa idrica, abbiamo la maggiore percentuale di perdite di un bene fondamentale qual è l'acqua e non utilizziamo le risorse per uno degli obiettivi previsti? È normale che non interveniamo sul fronte degli investimenti energetici? È normale che non mettiamo in campo investimenti su trasporto e mobilità sostenibile e per le imprese, così come indicato dalla Commissione europea?

anche a chi parlava di mancanza di esclusione delle infrastrutture): innanzi tutto, al comma 2 dell'articolo 11, si fa riferimento in modo molto chiaro allo sviluppo degli interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Perché dite che non c'è il tema infrastrutturale? È inserito nel decreto, al comma 2 dell'articolo 11, che parla della perequazione infrastrutturale. Il tema delle risorse è chiarito ancora meglio, perché se andiamo dietro alla polemica sull'importo

pluriennale degli investimenti, che al momento, nell'ambito del bilancio del nostro Paese, è pari a 6 miliardi di euro. Se si considera il 40 per cento di 6 miliardi, parliamo di 2,4 miliardi di euro per ogni annualità, quindi evidentemente non stiamo parlando di una scelta che penalizza, ma che mette a disposizione ulteriori risorse in questa direzione e rappresenta un'opportunità in coordinamento con le altre risorse che mettiamo in campo e anche e soprattutto con le scelte che vedono in questo decreto-legge anche altri aspetti molto importanti. Ho ascoltato anche critiche su alcune misure collegate, per esempio alle politiche del lavoro, sul tema degli *under* 35. Lo dico ai colleghi che le hanno sollevate: sono i programmi comunitari che danno queste indicazioni, non è una scelta del Governo. Noi in questo decreto-legge ci stiamo muovendo non dove vogliamo; stiamo rimodulando e compiendo scelte dentro la politica di coesione, che ha una programmazione europea di 43 miliardi di euro di risorse europee che diventano quasi 75 con il cofinanziamento nazionale e regionale, che si inserisce in una programmazione più ampia quale quella che abbiamo messo in campo e che per la prima volta mette in campo anche risposte concrete rispetto agli obiettivi per i quali dover realizzare finalmente gli interventi per i quali riceviamo queste risorse. Dobbiamo, infatti, dirci con chiarezza che che il meccanismo dei progetti sponda, cioè della possibilità di rendicontare progetti precedenti, ha portato a creare il cosiddetto concetto delle risorse liberate, risorse che vengono rendicontate per un intervento che non è stato realizzato con quelle modalità e che vengono utilizzate all'interno dei bilanci, soprattutto regionali, ma anche nazionali, in modo libero. Noi abbiamo creato un meccanismo per il quale, se prendi le risorse per quegli obiettivi, realizzi quegli obiettivi; e lo fai anche all'interno dei singoli programmi nazionali, nei quali noi non abbiamo compiuto scelte differenti. Abbiamo compiuto scelte che, dal punto di vista delle soluzioni settoriali sul mondo del lavoro, nell'ambito della ricerca, dell'università, delle infrastrutture, hanno una tempistica precisa e degli obiettivi chiari, che non possono essere in alcun modo essere messe in discussione. Noi, infatti, prendiamo queste risorse per fare questo, non per fare altro. Quindi, è inimmaginabile continuare a fare altro. Voglio anche cogliere l'occasione, visto che è stato sollevato il problema, per un chiarimento sul tema della decontribuzione e delle assunzioni al Sud. La Sud. La discussione è abbastanza particolare su questo tema. L'Italia non ha ottenuto una misura fino al 2029, come spesso sento raccontare; l'Italia ha presentato una misura che, nella sua legge nazionale, reca la previsione del 2029, ma che aveva bisogno di una notifica e di un'approvazione da parte della Commissione europea. Tale approvazione è stata data per sei mesi, al massimo per un anno, di volta in volta, sulla base del *temporary framework* per il Covid-19, cioè come misura straordinaria. Quando è scaduta, alla luce di quello che è successo con l'invasione dell'Ucraina, la misura è stata prorogata. Quando

ha ottenuto, con una complessa trattativa con la Commissione europea, è una proroga di altri sei mesi, che sono veramente straordinari, per i quali ho avuto modo, questa mattina a Bruxelles, di ringraziare la vice presidente della Commissione europea Margrethe Vestager, perché è con la sua direzione generale che abbiamo trattato questa proroga ulteriore di sei mesi sei mesi nei quali dobbiamo trattare una nuova misura di decontribuzione, differente da quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Non è possibile,

Concludo con una riflessione di carattere più generale. È stato citato, per una critica, lo Svimez. Io vorrei ricordare, non per assumere particolari meriti, ma come dato oggettivo, che, nonostante la discussione che si è tenuta su questo testo, non sono stati citati i dati dello Svimez usciti la scorsa settimana relativamente al Mezzogiorno d'Italia e all'anno 2023. In questi dati, c'è una crescita del prodotto interno lordo, a fronte di una media nazionale dello 0,9, dell'1,3 per cento nel Mezzogiorno. Non si tratta di assumersi nessun merito. Si tratta di prendere atto di un dato, di un dato, che è indicativo di come ci sia una politica che sta iniziando a dare delle risposte. Non è possibile, infatti, immaginare di attribuire responsabilità quando i dati sono negativi e di ignorare e non citare i dati quando sono positivi, come in questa circostanza.

in opere pubbliche, che cresce da 8,7 a 13 miliardi di euro. Sono dati che sicuramente rappresentano segnali positivi, un lavoro che va ancora implementato in questa direzione e che stiamo cercando di portare avanti con risultati che sono, dal nostro punto di vista, importanti e positivi, perché danno l'idea di una visione d'insieme che abbiamo messo in campo. Nella riorganizzazione complessiva dell'uso di queste risorse, infatti, noi stiamo affrontando un tema che lascia intendere che stiamo cambiando negativamente un sistema che precedentemente funzionava. Noi stiamo intervenendo sulla politica di coesione, cioè sulla parte delle risorse europee che rappresenta da sempre un elemento di grave preoccupazione, che ha creato un danno reputazionale al nostro Paese. È un dato oggettivo. Ho citato, all'inizio del mio intervento, il rapporto che la Commissione europea ha fatto sulla politica di coesione: l'ottavo rapporto nel 2022 e il nono del 2023. Basta leggere questi rapporti per capire la mancanza di efficacia di questa politica del nostro Paese e la necessità di intervenire in questa direzione. Il mio approccio è quindi quello di chiedere un lavoro comune su questo, non una valutazione critica a prescindere su elementi che spesso non troviamo all'interno di questo testo e soprattutto, laddove possibile, sarebbe auspicabile immaginare anche contributi che possano andare nella direzione di migliorare ulteriormente le scelte che andremo a fare. Nell'ambito del presente decreto-legge coesione, infatti, facciamo delle scelte che puntano ad accelerare la spesa di queste risorse, se è vero, come è vero, che questa programmazione ha la necessità e l'obbligo di spendere il 20 per cento dell'intero programma entro il 31 dicembre 2025; tuttavia siamo anche in una fase nella quale abbiamo la possibilità di aprire un confronto con la Commissione europea per rivedere le altre quattro annualità dopo il 2025. Questo è un tema molto importante, perché rivedere quelle priorità può voler dire anche individuare esigenze concrete che dovessero emergere e obiettivi che dobbiamo cercare di raggiungere. il nostro approccio è questo. Mi dispiace ascoltare alcune critiche sulla mancanza di visione, ma il punto forte della strategia del Governo Meloni su questo tema è proprio la visione, è proprio aver immaginato una visione completa, d'insieme delle scelte che abbiamo messo in campo anche e soprattutto rispetto a una capacità concreta di dare risposte settoriali rispetto alle letture messe in campo su questo terreno, sia nell'ambito degli strumenti che abbiamo predisposto, sia nell'ambito anche di altre scelte che sono coordinate, come per esempio quella sulla zona economica speciale. Al riguardo anche in questa sede ho ascoltato delle critiche, ma nei prossimi giorni presenterò in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento una relazione sul monitoraggio del lavoro delle otto zone economiche speciali per poter valutare la situazione che emerge da quell'esperienza e per poter anche dare una risposta ad alcune critiche che ho ascoltato rispetto alla inesistenza della struttura e alla mancanza di interventi. Tali rilievi, che non solo non corrisponde nemmeno lontanamente alla realtà dei fatti, ma soprattutto omettono un elemento un po' particolare, cioè che anche sulla ZES c'è una strategia collegata ad un altro elemento molto importante, che ha visto il Governo Meloni dare un'indicazione fondamentale per l'Italia, per il Sud Italia come centralità all'interno del Mediterraneo col Piano Mattei. Il fatto di aver creato una zona economica speciale al centro del Mediterraneo, che non riguarda otto piccole aree

possa svolgere un ruolo sempre più efficace in questa direzione e sempre più in grado di attrarre eventuali opportunità e nuovi investimenti. Tutto ciò ha il fine di creare le condizioni perché quella semplificazione dal punto di vista autorizzativo, le opportunità collegate agli incentivi fiscali e il piano di infrastrutturazione fondamentale in questa direzione possano costituire, proprio in questo ambito, in questa visione, una strategia d'insieme che completa il percorso che il Governo ha messo in campo

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento

lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; - l'articolo 15-*ter* sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.». Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1133, di conversione del decreto-legge 7 maggio n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60, nel testo proposto dalla Commissione, con le modifiche richieste nel parere espresso dalla 5a Commissione

Come il Ministro sa bene, abbiamo dato ampia disponibilità, su questo provvedimento, a ragionare di alcune eventuali, potenziali modifiche, proposte anche con nostri emendamenti e speravamo di poter fare una discussione anche in Aula. Ci sono 308 emendamenti che al Senato si esauriscono in qualche ora di votazioni, quindi non è chiaro perché anche oggi il Governo ponga la fiducia su un provvedimento che, con il contributo del Senato, avrebbe potuto avere un miglioramento. Fermo restando che, come ho detto in Commissione, avendo seguito il provvedimento - lo ricorda probabilmente il Ministro - alcuni spunti di questo provvedimento erano condivisibili e avrebbero potuto vedere la compartecipazione della mia forza politica anche in ottica di un voto non per forza negativo. È chiaro che con la fiducia tutto questo salta e ci dispiace che venga umiliata la possibilità del Senato di contribuire al miglioramento di un testo che poteva

l'ampio confronto e soprattutto la disponibilità del Partito Democratico ad essere propositivo e costruttivo, non abbiamo fatto ostruzionismo.

Non si rafforza in questo modo il ruolo del Parlamento. Sarebbe invece stato molto interessante interloquire con il Ministro, in particolare dopo le sue repliche, che contengono anche tante cose inesatte sbagliate, perché la programmazione dei fondi di sviluppo e coesione era già regolata anche nella legislatura precedente, con patti che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni. ha parlato del fatto che questo Governo ha una sua visione, ma francamente la visione dello sviluppo economico e sociale di questo Governo, su come il Paese si prepara ad affrontare un nuovo modello di sviluppo, per quello che ci riguarda è incomprensibile e assente, quindi questo è un Governo senza visione e ci sarebbe piaciuto molto in quest'Aula poter interloquire con gli emendamenti evidenziando anche le nostre proposte, cosa che il Governo, ponendo la fiducia, ha voluto evitare. Quindi, se fosse possibile, anche noi gradiremmo poter discutere questo provvedimento senza l'ennesima fiducia, che è un colpo mortale al Parlamento e al ruolo di quest'Assemblea.

Noi, insieme ai colleghi che mi hanno preceduta, in Commissione bilancio abbiamo lavorato in uno spirito costruttivo. Pensi, signor Ministro, che solo oggi sono arrivate tre corpose modifiche per una serie di errori che sono stati commessi nel corso della costruzione del provvedimento; anziché fare le barricate, metterci a fare delle riunioni fiume in Commissione, abbiamo rispettato l'ulteriore implementazione di correzioni che sono state fatte nel corso di tutto il provvedimento. A fronte di ciò, abbiamo presentato emendamenti del tutto ragionevoli e abbiamo condotto una discussione in un clima di serietà e, anche con anche con il presidente Calandrini, sempre di collaborazione. Tutto mi sarei aspettata tranne che il voto di fiducia su un provvedimento che poteva avere

Come il segnale di un po' di stanchezza di questa maggioranza? Un conto è mettere la fiducia su questioni sulle quali ci sono dei problemi oggettivi dal punto di vista politico. Però, se fate così sul decreto-legge coesione, cosa farete quando invece si tratterà di votare provvedimenti ben più complessi dal punto di vista finanziario? Non lo so. Ripeto e dico in maniera è il frutto di un po' di difficoltà che ci sono e che francamente, secondo me, non risolverete in questo modo. Ve lo dico con franchezza. Peccato, perché dentro questo provvedimento potevano esserci anche dei punti votabili; però, se a voi non interessa che ci sia una collaborazione dentro il Parlamento, sarà quel che sarà, cioè sarà una discussione ideologica e dogmatica. Non so dove vi porterà, ma secondo me vi porterà

indipendentemente dalle valutazioni che ognuno di noi fa, abbiamo anche ridotto il numero degli emendamenti per l'Aula. Ognuno di noi ha cercato di autoregolarsi e di arrivare in Aula

con cui contribuire, purché ci si ascolti. Invece il dato fondamentale è un'arroganza da un certo punto di vista. La cosa che più mi preoccupa è svilire i

il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con modifiche e integrazioni, reca un complesso di modifiche normative in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. L'articolo 1 estende alle forme associative dei Comuni, ivi comprese le Comunità montane, isolane e di arcipelago, la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali vigenti. Le assunzioni in oggetto, effettuate dalle forme associative comunali, così come già previste per quelle suddette dei singoli Comuni, devono avvenire nell'ambito delle risorse richiamate dall'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni. Resta fermo il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio. Il comma 1 dell'articolo 2, novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e successive modificazioni, istituisce, nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate e finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie. Per la partecipazione al tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo o suo delegato presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte

concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori. In particolare, la novella introduce in via aggiuntiva la previsione di una relazione annuale specifica concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori. L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. L'istituzione di tale giornata è intesa ad informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione al diritto del medesimo. Si prevede che, ai fini della celebrazione della Giornata, le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado realizzare campagne pubblicitarie nazionali di carattere sociale. Il comma 3 specifica che la Giornata non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. L'articolo 4, che consta di un unico comma, reca alcune modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del luglio 2017. La lettera *a)* specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivati dai rapporti di sponsorizzazione promo-pubblicitari, concessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. La successiva lettera *b)* prevede, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. in primo luogo modifica la disciplina sulla possibilità di attuazione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Le modifiche, tra l'altro, elevano il limite nella misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto del nuovo limite più basso, la possibilità

lettera *m)* modifica l'articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore e successive modificazioni; comma concernente la possibilità, relativamente alle attività diverse da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera Grazie, ci consente in via ordinaria, salvo divieto espresso all'atto costitutivo nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'indennità dell'associato che partecipi ai voti. Le lettere *e)* e *f)* recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore e successive modificazioni, con riferimento rispettivamente alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non riconosciute nel Terzo settore e alle ipotesi che determinino l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime. La lettera *g)* modifica l'articolo 36 del codice del Terzo settore, settore, relativo ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale. La lettera *h)* inserisce il comma 2-*bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislativa e deve essere integrato entro un anno. Le lettere *i)* e *l)* modificano gli articoli 47 e 48 del codice del Terzo settore. Le novelle concernono la domanda d'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore. La lettera *n)* prevede la possibilità di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari di categorie in congedo.

Italia sociale. Si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione sia estinta e liquidata. L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale agli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile.

Signora Presidente, ringrazio la relatrice e i membri di Commissione per i contributi che hanno dato e anche per gli altri approfondimenti che sono stati svolti attraverso le audizioni. È un disegno di legge che tende a dare risposte alle politiche sociali, ai più fragili, in particolare ai minori senza famiglia, ma anche al Terzo settore, con un pacchetto di prime semplificazioni, nella gestione amministrativa e burocratica, sciogliendo alcuni nodi che sono rimasti insoluti rispetto al codice del Terzo settore che è stato inaugurato nel 2017. È un primo pacchetto di riforma al quale faranno seguito altri, collazionato con tutti i protagonisti: gli enti del Terzo settore, in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore, ma anche al Forum del terzo settore. Quindi, è un lavoro corale con le categorie di rappresentanza, i notai, gli avvocati e i commercialisti, tutti coloro che hanno contribuito a inserire delle norme di buonsenso.

mi scuso se la voce è fioca, ma a detta dei medici ho straviziato un po'. Ora, a una persona cosiddetta normale, se fa un aperitivo al giorno morigeratamente, si dice "bravo"; quando però la stessa cosa la fa una persona con disabilità allora stravizia: evidentemente, il giudizio implica una disabilità o la normalità, per cui quello che si vive nella normalità è tutto normale, mentre quello che si vive con disabilità sembra vizioso. Sono molto orgoglioso dei miei vizi, che non fanno male a nessuno, almeno credo, ma toccherebbe chiederlo a chi mi ama. Sono molto sereno nel rappresentare questo provvedimento che, per motivi anche…

Fa parte della mia vita il Terzo settore. Ricordo con nostalgia - mi venga permessa - quando, decenni fa, ad Assisi,

insiste nel fare - parlai del Terzo settore come della colonna vertebrale del nostro Paese. Dico che oggi è ancora più vero. In questo periodo così complesso, il Terzo settore è

l'apertura che il Governo fa. Tra l'altro, mi sono molto rasserenato nel sentire per l'ennesima volta Raffaele Fitto, con la sua calma, con la sua scientificità politica e il suo rispetto per la maggioranza e l'opposizione, dire che non ha visione. Come ha detto il senatore Misiani, significa significa non saper leggere. Qualche analfabetismo lo perdoniamo ancora. La lungimiranza del Governo, per quanto mi riguarda, mi gratifica due volte: per l'attenzione, nuova e più concreta, al Terzo settore, ma anche per l'apertura nuova, detta, esplicitata all'infanzia, all'adolescenza e a quel periodo, così particolare,

che ha sempre visto in modo problematico gli assistenti sociali, ne parla bene. Ci mancherebbe altro: io ho sempre lavorato con le assistenti sociali che, pur essendo capo servizio, non ho mai definito mie. Però, qualche volta, in assenza di un famiglia, ma anche di una realtà di ascolto reale per la famiglia lo so perché l'ho fatto e bisogna tradurlo in realtà locali - è molto difficile che l'infanzia venga ascoltata. E lì, forse, il potere di molte, troppe assistenti sociali

delle differenze territoriali che, in un'unica azione, vengono esaltate e non cancellate. Poi esiste la Commissione, che si estende all'infanzia e all'adolescenza, ma soprattutto al periodo così fluido

fase della vita di una persona, così delicata, forse non recepiremo più una voglia di vivere, una voglia di autorappresentarsi, che non deve essere mai demonizzata, mai miticizzata, mai esorcizzata. Bisogna tenerne conto, con un po' di umiltà. Forse, quando si applicano provvedimenti così delicati, ci vuole scientificità, ci vuole amore per la politica, ci vuole anche un po' di umiltà. Ne sappiamo qualcosa, avendo gestito, oltre che la politica, anche associazioni così delicate. Vi è poi il discorso dei finanziamenti, il fatto di tener conto di realtà che finora non sono state addirittura prese in considerazione, delegando tutto ad associazioni un po' di bandiera o di sindacato. Concludo - anche perché la voce mi assiste poco che qualche volta si può dare un parere positivo anche sull'onda del consenso del consenso del proprio partito, della propria coalizione, del proprio Gruppo; questa volta, proprio per motivi prima di tutto professionali e poi politico-partitici, esprimo un parere estremamente favorevole e, se mi fosse permesso di dirlo, Abbiamo bisogno di entusiasmo, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno - perché no? - di dare a chi vive la politica dall'esterno, ma poi in realtà tutti fanno politica anche quando dicono che sono disinteressati e non votano (anche quella è una politica). Bisogna dar loro speranza e questo provvedimento dà una speranza che diventerà senza dubbio concretezza.

su questi temi che riguardano provvedimenti così importanti come le politiche sociali e la riforma del Terzo settore, da sempre da sempre come Italia Viva vorremmo lanciare un messaggio positivo. Crediamo che su questi temi bisognerebbe avere avere un'ampia maggioranza e soprattutto un confronto, che c'è stato su molte questioni e su molti temi. D'altra parte, condividiamo gran parte dei contenuti del testo anche nella direzione di una certa continuità con la grande riforma del Governo Renzi proprio sui temi che riguardano le politiche sociali e il Terzo settore. Mi fa piacere poter dire anche in questa sede che, nonostante l'alternanza dei Governi, c'è stata una certa continuità su alcune questioni; su altre, però, la direzione non è stata proprio questa, a cominciare dal tema delle risorse. Noi sappiamo che anche i dati di qualche giorno fa dell'Istat ci dicono purtroppo che la povertà continua ad aumentare

piccoli - nelle attività quotidiane, nel dare risposte ai loro cittadini, alle famiglie che sono sempre più povere.

di aiutare le tante marginalità oggi presenti nei nostri territori. Noi avevamo chiesto di istituire un fondo da 40 milioni di euro per aiutare i Comuni nella presa in carico non solo delle varie marginalità, ma soprattutto sulla questione che riguarda i minori, perché sappiamo che la povertà minorile e il disagio giovanile sono dei grandi problemi in continuo aumento. Su questo avremmo preferito più concretezza e meno slogan; avremmo preferito meno giornate del ricordo e invece più risorse adeguate per gli amministratori di tutti i colori politici, ovviamente. Va benissimo, certamente, aver istituito la Giornata dell'ascolto dei minori, ci mancherebbe. Tuttavia, signora Vice Ministra, anche se so che lei ha una grande sensibilità su questi temi, dobbiamo coinvolgere certamente tutto il mondo delle scuole, il personale, le tantissime professionalità, le competenze di cui è ricco il nostro Paese. Abbiamo bisogno, insomma, di guardare alla riforma del Terzo settore in maniera molto più strategica per i prossimi mesi e, d'altra parte, chi fa una riforma deve avere una visione del Paese almeno da qui ai prossimi dieci anni. Su questo vorremmo che ci fosse un coinvolgimento ancora maggiore di tutti gli attori, di tutti i protagonisti che abbiamo nei territori: quindi una maggiore coesione territoriale, servizi socioassistenziali riparativi, cultura, agricoltura sociale, sport, formazione professionale, tutti temi che devono riguardare questa grande riforma e il codice del Terzo settore.

sport. È importante che gli enti sportivi dilettantistici si iscrivano anche al Registro unico nazionale del Terzo settore per poter beneficiare delle stesse opportunità. Penso, ad esempio, al tema del cinque per mille, al tema delle donazioni, del *social bonus*,

Il nostro partito ha presentato un disegno di legge anche a tal riguardo, che chiede stabilità, per esempio, sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni territoriali. Sarebbe un modo pulito e trasparente per aiutare le società sportive dilettantistiche e e quegli imprenditori che vogliono sponsorizzare la propria squadra, la propria associazione di riferimento. Questo non possiamo più legarlo a una finanziaria o all'altra, sapendo che le risorse sono sempre meno e sarebbe necessario, quindi, avere un fondo *ad hoc* anche per questo. Consideriamo molto positiva poi la misura di coordinamento rispetto ai bilanci, perché sappiamo che gli enti sono diversi - gli enti di formazione, gli enti che si occupano di istruzione - e giustamente tengono in conto di avere anche un esercizio diverso rispetto agli altri. Consideriamo positiva la norma sulle ONLUS che, proprio perché prevalentemente a partecipazione pubblica, non entreranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ad esempio, bisogna accelerare sulle misure di favore rispetto alla fiscalità del Terzo settore, perché è importante che in questa fase tutti possano essere aiutati allo stesso modo. modo. Credo che su questo bisognerà lavorare ancora molto, perché il Terzo settore - lo sappiamo - ha tante sfaccettature, ma ricordo - perché i numeri sono importanti - che oggi ci sono 5,5 milioni di volontari che sono una parte fondamentale del nostro Paese, insieme a quasi un milione di lavoratori e di lavoratrici che operano nel settore. settore. Dobbiamo vedere il Terzo settore come un'economia sociale, un motore di sviluppo, una competenza europea e ciò significa investire non soltanto sul significato etico che oggi ha il volontariato, ma anche sulle professionalità e sulle competenze. Se ne parla tanto, ma poi sappiamo che molti enti, molte associazioni invece non ce l'hanno fatta e hanno dovuto chiudere e sono migliaia sui nostri territori e spesso sono l'unica gamba, l'unico strumento che può dare a quella comunità un aiuto, un *(Applausi)*. C'è poi un altro aspetto. Voi sapete che la posizione di Italia Viva sul *bonus* 110 è molto chiara e lo è sempre stata fin dall'inizio. È un'eredità negativa, è stata lasciata sulle spalle dei cittadini e delle imprese, ma c'è un punto: non possiamo permetterci di far fallire tante realtà sociosanitarie e socioassistenziali che, peraltro, sono state inserite nelle opportunità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Termino dicendo che dobbiamo aiutare soprattutto le associazioni e gli enti: penso anche alle RSA e a tutti coloro che fanno un lavoro magari invisibile, perché basato su tanto volontariato, ma molto utile al nostro Paese. Mi auguro che questa riforma abbia davvero le gambe per poter camminare in maniera celere, ma soprattutto abbia le risorse necessarie per dare stabilità ad un quadro del Paese che vede sempre di più crescere un divario sociale e culturale molto preoccupante, soprattutto se guardiamo alla povertà minorile. Per tutte queste ragioni, signora Presidente, il voto di Italia Viva sarà di astensione.

che ha introdotto un elemento importante sul terreno del Terzo settore. Il terzo settore è diventato sempre più pesante

del 2016, con i decreti attuativi, ha appesantito in alcuni comparti del Terzo settore la burocrazia, con il rischio che alcuni servizi vengano meno.

Abbiamo visto anche appesantirsi molto la regolamentazione. Eppure questo settore produce circa il 5 per cento del PIL nel nostro Paese, perché dà

la socialità. Ad esempio, durante il Covid molte attività del Terzo settore hanno rischiato di saltare dal punto di vista dell'attività sociale;

forse bisogna porsi il problema di come si finanzia un elemento. Abbiamo parlato prima del decreto coesione, ma anche la socialità, anche il fatto di avere un terzo settore che funziona è un elemento di coesione, un elemento di coesione e socialità per tutta la società, quindi è un bene. Però allora bisogna spendere risorse in questa direzione e a noi non pare che ci siano risorse a sufficienza.

sia perché c'è già la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia perché, francamente, non si avverte la necessità necessità di istituire un'ulteriore giornata. Ci sarebbe bisogno di ulteriori interventi ben finanziati, tenuto conto del livello di risorse molto al di sotto delle necessità. Per questa ragione - l'ho fatta molto breve

Grazie, Presidente. Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, il disegno di legge al nostro esame è stato esaminato in sede redigente dalla 10a Commissione del Senato, che ha approvato il testo senza modifiche, pur avendo approfondito le tematiche con ulteriori audizioni. Il disegno di legge di iniziativa del Governo contiene modifiche puntuali al codice del terzo settore, che sono state apprezzate innanzitutto dagli stessi operatori del terzo settore, nuovamente auditi qui in Senato. La Camera ha aggiunto ulteriori articoli che hanno completato e arricchito il complesso dell'articolato. Ecco perché ci sentiamo di condividere un testo che segna un passo in avanti in favore di chi opera nell'interesse degli altri e lo fa ogni giorno, con un impegno e con servizi che spesso vanno a integrare quelli offerti dalle strutture pubbliche. Si interviene con norme da loro stessi richieste e che migliorano le modalità e gli spazi in cui intervengono gli operatori del sociale a favore dei cittadini. Innanzitutto vengono modificate e integrate le norme del codice del terzo settore, adeguandole al nuovo contesto emerso dopo gli anni della pandemia. Viene ampliata la possibilità, per gli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, di scrivere il bilancio in forma semplificata. Sono presenti inoltre disposizioni che puntualizzano il rapporto delle associazioni sportive dilettantistiche con le sponsorizzazioni, consentendone l'utilizzo per attività di interesse generale. Vengono alzati i limiti per i quali le associazioni debbono nominare un revisore legale. Inoltre, viene alzata la percentuale di lavoratori rispetto a quella degli associati, per poter impiegare forza lavoro nell'associazione di promozione sociale. Sono state modificate anche le disposizioni del RUNTS, il Registro unico nazionale del terzo settore, per semplificarne l'accesso ai dati con nuove norme anche per l'approvazione e il deposito dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS e presso il registro delle imprese. La possibilità di iscrivere al RUNTS le associazioni di militari in congedo e pensionati che svolgono determinate attività di interesse generale è un altro elemento da valutare con assoluto favore. Insomma, il complesso delle modifiche e delle nuove norme introdotte rappresenta un presidio essenziale, a tutela dell'attività associativa senza scopo di lucro. Quindi, si tratta di semplificazioni amministrative e disposizioni per un più puntuale reperimento delle risorse necessarie a far funzionare l'articolata macchina della solidarietà sociale. È apprezzabile anche l'estensione per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, comprese le Comunità montane e quelle isolane. Sappiamo quanto sia importante il ruolo svolto da questi lavoratori nelle nostre comunità, per cui le disposizioni previste sono da accogliere positivamente. La Camera ha voluto introdurre un tavolo nazionale per l'inclusione sociale dei minori fuori famiglia, di quelli in affido e in carico ai servizi sociali: un tema delicatissimo che riguarda i soggetti più vulnerabili, che vedrà il coordinamento e il monitoraggio degli interventi da adottare a tutela di queste categorie fragili, ma che vedrà coinvolto anche il lavoro della Commissione infanzia, che sarà relazionata dal lavoro del tavolo e della rete per la protezione e l'inclusione sociale. A favore di una maggiore sensibilizzazione, ogni 9 aprile ci sarà la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, per la quale le scuole potranno promuovere apposite iniziative di coinvolgimento delle comunità scolastiche. L'inclusione dei minori è uno dei temi fondanti di qualsiasi società che voglia definirsi civile e inclusiva e queste disposizioni vanno proprio nella direzione di adottare interventi di maggiore inclusione e protezione nei confronti dei minori che non hanno una famiglia che li possa seguire. Va ricordato come molte norme concrete di questo Governo - mi riferisco, ad esempio, a quella del cosiddetto decreto Caivano - sono già andate in questo senso, riguardando non solo la realtà di Caivano, ma tutte quelle aree nazionali in cui avviene l'esposizione dei minori al degrado e all'emarginazione. Quindi, siamo in presenza di un complesso di disposizioni destinate a sostenere gli ambiti dell'inclusione e del sociale, che opera a sostegno dei cittadini, spesso degli ultimi della società, all'insegna della piena solidarietà. Vorrei concludere questa dichiarazione di voto, che ovviamente vede favorevoli i senatori di Forza Italia, con il ricordo di Claudia Fiaschi,

rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è un disegno di legge di iniziativa del Governo recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore, che, con il lavoro emendativo svolto alla Camera anche dal nostro Gruppo politico, MoVimento 5 Stelle, è stato trasformato fino a diventare una sorta di piccola riforma del codice del terzo settore. Nell'ambito di questa piccola riforma, riconosciamo alcuni aspetti positivi che apprezziamo, mentre per altri osserviamo criticità, che evidenzierò nel corso del mio intervento. Condividiamo la previsione di un aumento degli assistenti sociali sul territorio, avendo però attenzione maggiore rispetto ad una loro specifica professionalità e formazione. Su tali aspetti, purtroppo, si è assistito sempre di più ad una standardizzazione dei servizi a discapito del benessere del minore e delle famiglie. Pertanto, sarebbe auspicabile che, oltre all'aumento numerico degli assistenti sociali, ci fosse anche una preparazione e una consapevolezza da parte degli operatori che devono svolgere le loro attività nell'unico interesse dei soggetti fragili. Inoltre, troviamo critiche le modifiche che hanno innalzato la soglia limite oltre la quale diventa obbligatorio, per le associazioni riconosciute e non riconosciute del terzo settore, nominare un organo di controllo contabile e un revisore legale dei conti. Il rischio è che, nel tentativo di semplificare il sistema di gestione del terzo settore, si vadano poi ad inficiare i meccanismi di controllo, di trasparenza e gli opportuni sistemi di tutela. Con riferimento poi alla distribuzione del numero di assistenti sociali, la gran parte delle Regioni ha una ripartizione meno uniforme, con aree ben strutturate e altre gravemente deficitarie.

ha prodotto un numero di 1.688 assistenti sociali. Si tratta di un numero che non riteniamo molto elevato e complessivamente non sufficiente, soprattutto a coprire le evidenti sperequazioni che esistono tra i territori.

È cresciuto in queste Regioni, ma in quelle del Mezzogiorno il rapporto tra assistenti sociali e abitanti resta inferiore al livello essenziale, quindi di gran lunga inferiore al rapporto di 1 a 5.000 abitanti introdotto grazie all'approvazione di una nostra proposta emendativa.

Oggi ci attendiamo da questa maggioranza che venga raggiunto un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, tutto ciò per potenziare ulteriormente il sistema dei servizi sociali comunali e per renderli uniformi su tutto il territorio nazionale. Veniamo ora al capitolo delle risorse: quelle con cui finanziare le assunzioni sono relative a due diversi fondi distribuiti ai Comuni, la quota parte del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, innanzi tutto, e poi la quota parte del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali. Apprezziamo l'articolo 2 del provvedimento, con il quale viene istituito un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e dei minori affidati in carico ai servizi sociali territoriali. Tuttavia, reputiamo opportuno prevedere, tra gli otto rappresentanti di organismi del terzo settore partecipanti al tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, la presenza di un membro facente parte di associazioni di persone con disabilità di rilievo nazionale, quale portatore di interessi e dei bisogni dei minori con disabilità. Ci dispiace molto, signor Vice Ministro, che un emendamento che andava in questa direzione non sia stato accolto da questa maggioranza, evidentemente sorda alle richieste fatte dalle associazioni di categoria delle persone con disabilità. Non contesto il principio di base che vede proprio nell'informazione e nella conoscenza il presupposto fondamentale per dare concretezza e attuazione ai diritti dei minori, ma mi risulta difficile pensare e immaginare che, istituendo una giornata senza prevedere coperture (nessuna copertura), sempre a invarianza di spesa, come tutto questo decreto, si riesca in qualche modo a raggiungere l'obiettivo. Senza risorse, si rende di fatto questa giornata una misura puramente simbolica. Ora però arriviamo alla nota che duole: questo disegno di legge puntualizza che la norma si possa tradurre in azioni concrete a costo zero, ovvero possa avvenire fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (sostanzialmente, quindi, a invarianza finanziaria), mentre per noi era necessario prevedere un maggior investimento di risorse anche e soprattutto per monitorare il meccanismo di spesa e formare il personale necessario all'accesso ai fondi. È questa una delle tante urgenze che questo Governo avrebbe potuto affrontare, se non fosse per il fatto che avete deciso invece di rinunciare ai tre miliardi di extraprofitti bancari o di dare priorità a progetti come il ponte sullo Stretto di Messina, destinandovi 14 miliardi. Ormai è chiaro agli italiani che, quando si tratta di destinare fondi per aiutare le persone più fragili, chiudete le orecchie e gli occhi e vi girate dall'altra parte, dalla parte dei più forti e dalla parte dei poteri forti. In considerazione di ciò, il MoVimento 5 Stelle si asterrà. Signor Presidente, vorrei iniziare dicendo grazie: grazie alle tante associazioni ed enti del terzo settore che esistono in Italia; grazie ai tanti volontari, circa quattro milioni e mezzo, che, nella loro attività quotidiana e gratuita, garantiscono quei servizi necessari ed essenziali che il nostro sistema pubblico non riesce a garantire completamente. Un settore che diventa indispensabile per la quotidianità e per il *welfare* sociale; un settore che ha dimostrato di esserci sempre, nella quotidianità, per anziani e disabili, per i fragili, ma anche nelle grandi catastrofi naturali, come i terremoti, scavando ad Amatrice e a L'Aquila, o con le mani nel fango, come nelle diverse alluvioni avvenute purtroppo in diverse Regioni, come per esempio l'Emilia-Romagna da cui provengo, di questi giorni, in cui ci sono stati problemi in diversi territori. Non dimentichiamo quello che hanno fatto silenziosamente questi enti ed associazioni durante la pandemia. Grazie a tutti. Il terzo settore è una realtà da sostenere e rilanciare. Ecco perché la riforma adottata nel 2017 attendeva di essere completamente attuata. Ed ecco perché questo Governo ha voluto dare una risposta concreta, sistemando quelle criticità e storture che aspettavano da tempo. Si tratta di un lavoro che era iniziato con la legge di bilancio che, ad esempio, ha semplificato e uniformato le modalità di monitoraggio, ma anche di rendicontazione, del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, grazie alla ministra Erika Stefani e adesso alla ministra Locatelli. Tale lavoro ha anche derogato al tetto per l'assunzione da parte degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome, relativamente alla gestione del registro unico familiare degli enti del terzo settore. Il percorso è proseguito con questo disegno di legge che ci accingiamo a votare, fatto dell'ascolto attento dato da questo Governo al mondo del terzo settore, che chiedeva di semplificare, di rivedere la parte burocratica ed amministrativa. perché, con l'entrata in vigore del codice, molte associazioni ed enti di volontariato hanno dovuto fare i conti con una serie di adempimenti e procedure burocratiche che hanno rallentato e complicato l'attività quotidiana, rischiando di compromettere le loro funzioni sociali. Ecco perché in questo disegno di legge viene estesa alle forme associative dei Comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale. Non solo: nell'ambito della rete dell'inclusione e della protezione sociale, viene istituito il tavolo nazionale di lavoro sui minori affidati ed in carico ai servizi sociali e territoriali e sui neo maggiorenni in prosieguo amministrativo. Questo tavolo, oltre ad essere formato dai Ministri e dai funzionari, intende anche avere la partecipazione di un rappresentante delle associazioni familiari tra le più rappresentative e di otto rappresentanti di enti del terzo settore. Questo è un segnale molto importante. L'articolo 3 istituisce nell'8 aprile la Giornata di ascolto dei minori, che ovviamente non ha effetti civili sulle festività e, come sempre, si celebrerà senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Negli articoli successivi vengono riviste alcune norme del codice del terzo settore. È modificata la norma specificatamente dedicata alle attività sportive dilettantistiche e quella sulle imprese sociali costituite in forma di associazioni e fondazioni. Si modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; si consente in via ordinaria la possibilità per i soci di intervenire utilizzando i mezzi delle telecomunicazioni e il voto per via elettronica. Si è aggiunto anche un altro emendamento del Governo, una novità importante, in favore delle associazioni d'Arma, che pone un rimedio ai problemi che si erano creati nel 2017 con la riforma del codice del terzo settore

Signor Presidente, la Lega crede fortemente nell'attività di volontariato come sistema solidaristico, indispensabile per la tenuta del nostro *welfare* sociale e pilastro importante del nostro sistema Paese. Un modello tutto italiano, che molti Paesi ci invidiano e che, grazie al ministro Locatelli, stiamo facendo conoscere a livello internazionale, con la sua partecipazione all'ONU oppure nell'organizzazione del G7, a ottobre in Umbria. Con questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega.

sarà capitato a molti di noi di riflettere su come sarebbe possibile essere comunità senza le attività, i presidi e servizi offerti dal terzo settore, una risorsa imprescindibile, che è davvero un vanto per il nostro Paese. Si tratta di un ambito indispensabile, stratificato e significativo, una rete preziosa, attiva da decenni e riconosciuta solamente in tempi recenti grazie a un Governo di centrosinistra. Sono certamente organizzazioni diverse per dimensioni e per tipo di attività svolta, ma tutte rispondono ai bisogni della comunità per il solo bene comune. Vogliamo essere chiari: per noi il terzo settore è una realtà da sostenere lavorando in sinergia con i territori. In questo modo ha promosso un profondo cambiamento sociale, che ha migliorato la qualità della nostra vita. I numeri lo confermano: l'aumento del 52,8 per cento di associazioni afferenti negli ultimi dieci anni e i 4,5 milioni di volontari stimati sono dati che raccontano di un settore in crescita, a indicare, dunque, la necessità sempre più forte di integrare e di supportare le istituzioni rispetto a nuove povertà, a solitudini emergenti, alle fragilità, alla carenza dei servizi. Solo per fare alcuni esempi, parliamo di un mondo che lavora nelle carceri per il reinserimento dei detenuti, con i migranti, con le persone con disabilità e fragilità. un settore che si è occupato del soccorso e della ricostruzione dopo le grandi tragedie naturali, che si impegna ad avere un Paese libero dalle mafie e dai ricatti quotidiani della criminalità organizzata; che non lascia soli gli anziani, che si oppone al razzismo e all'intolleranza, che aiuta le donne vittime di violenza, che lotta contro la dispersione e l'abbandono scolastico nelle realtà più marginali del Paese. Presidente, per essere davvero comunità, serve ridurre le diseguaglianze e certamente in questo il terzo settore svolge un ruolo determinante. Mi sembrava una premessa importante e desidero anche sottolineare che noi non siamo affezionati alle nostre riforme; siamo consapevoli che sia necessario rivedere ed aggiornare le norme per migliorare la risposta dello Stato. Tuttavia, nel caso di questo provvedimento il giudizio non è del tutto positivo: in sintesi, qualche novità positiva, ma tante ombre e tante soluzioni rinviate. Ben venga, dunque, l'ascolto attento dato al mondo del terzo settore, che chiedeva di semplificare e di rivedere la parte burocratico-amministrativa. È corretto avere esteso alle forme associative dei Comuni la possibilità di assumere a tempo indeterminato assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa, sebbene le risorse stanziate non siano comunque sufficienti. Tuttavia di questo hanno parlato i miei colleghi che mi hanno preceduto. Giungendo alle dolenti note, invece, ci lascia molto perplessi la norma che istituisce un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e dei minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e la previsione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei minori fuori famiglia.

il compito di monitorare eventuali anomalie e promuovere ispezioni. Qual è la ragione di questa duplicazione? Sembra quasi che ogni Ministero lavori senza alcun accordo su progettualità sovrapposte che creano confusione.

e proteggerli, perché i dubbi onestamente non mancano e con le vostre azioni rischiate di aumentare la confusione. Che dire, poi, della proposta di istituire il 9 aprile di ogni anno la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori? Non servono nuove giornate, mere bandierine di propaganda fine a se stessa, volte a intortare l'opinione pubblica. Servono risorse adeguate. Per noi la partecipazione è molto di più di una giornata di ascolto: è sviluppare il protagonismo dei nostri giovani, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, anche in attuazione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. In generale, signora Presidente, non sembra proprio che questo Governo si sia occupato realmente, oltre agli *slogan*, di minori. Il decreto immigrazione ha fatto saltare un pilastro di civiltà con il diritto alla protezione degli *under* 18; il decreto Caivano punisce per educare; oppure vogliamo parlare dei 210 euro di assegno restituiti dalle famiglie monogenitoriali o dei tagli agli asili nido, dello stop dell'IVA al 5 per cento per i prodotti per l'infanzia o ancora del taglio per i centri estivi? Ma è questa la coerenza del Governo? Non ci ingannate: difendere la famiglia significa riconoscere il lavoro di cura, ma anche riconoscere le professionalità come quelle degli educatori che ogni giorno assistono anziani, soggetti fragili, disabili, soggetti svantaggiati. Come Partito Democratico, porteremo sempre avanti tutte le battaglie per i diritti, la qualità della vita e la dignità delle persone. Ci troverete pronti quando verrà il momento di ricostruire i supporti alle nostre comunità, ai giovani, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà e che non riescono nemmeno più a curarsi. Non c'è futuro senza assicurare a tutte e a tutti istruzione, cure sanitarie, abitazioni dignitose, assistenza, previdenza pensionistica, sostegno al lavoro. Si poteva fare di più con questo disegno di legge, ad esempio accettando anche le proposte che abbiamo avanzato in Commissione e con gli emendamenti, dopo un percorso di ascolto delle realtà associative. La volontà di non modificare il testo per evitare il rinvio alla Camera blocca un percorso di riforma riforma necessario per dare risposte che gli enti del terzo settore chiedono da molti anni. È sintomatica la vicenda dei lasciti testamentari, che aveva visto adesione anche dal Ministero, che però non è stata accolta in questo testo. Occorre infatti completare la semplificazione normativa necessaria a sgravare gli enti da un appesantimento burocratico che comporta spesso ingenti spese e il ricorso alle vie legali prima di entrare in possesso dei beni. Un'occasione persa, così come l'emendamento per rafforzare la trasparenza delle modalità di utilizzo del cinque per mille da parte degli enti *non profit*, rafforzando il dialogo con i loro donatori e una richiesta che arriva dal terzo settore che non avete voluto accogliere per il desiderio di fare presto e portare a casa una legge senza pensare alle soluzioni che in questo modo perdiamo per strada. Per risparmiare il tempo della terza lettura si rinviano *sine die* norme che potevano essere tranquillamente inserite in questa seconda lettura al Senato. Con queste osservazioni ho provato a spiegarvi l'amarezza che rimane per un lavoro parlamentare che, alla fine, risulta essere frettoloso, impreciso, incapace di includere tutte le soluzioni ai problemi che in questi anni le realtà del terzo settore hanno portato alla nostra attenzione. nostra attenzione. L'Italia può dirsi fortunata, grazie al contributo fondamentale di associazioni e di organizzazioni della società che affiancano e spesso suppliscono alle carenze dello Stato, un contributo da valorizzare e mai impoverire, che meritava un impegno maggiore in quest'Aula. Per questi motivi, solo sintesi di molte altre perplessità che rimangono su questo provvedimento, annuncio il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, per prima cosa vorrei anch'io esprimere un sincero ringraziamento al vice ministro Bellucci per la passione, la competenza e la determinazione che ha posto in tutte le occasioni di discussione di questo provvedimento. alla relatrice Mancini e a tutti i colleghi e colleghe per il lavoro svolto in 10a Commissione. Il provvedimento che ci accingiamo a votare, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore. Si tratta di un intervento normativo importante e molto atteso, che interessa non solo specifici enti, ma ridisegna un settore, quello del volontariato nazionale, che a partire dagli anni Ottanta ha assunto un ruolo decisivo e un valore economico, sociale e culturale sempre più riconosciuto e apprezzato, come un volano di supporto in un settore, quello delle politiche sociali, che ha un ruolo strategico all'interno del tessuto connettivo della nostra Nazione. Ricordo anche il contesto temporale nel quale si inserisce, dopo gli eventi tragici della pandemia che ha portato a restrizioni mai viste della nostra libertà, con conseguenze radicali su tutto il nostro vivere la socialità. È proprio da quella drammatica esperienza che deriva non solo l'esigenza di riscrivere un modello sociosanitario che possa essere in grado di affrontare queste emergenze per il futuro, ma anche la necessità di recuperare ogni spazio per una sana vita sociale e recuperare quelle certezze nelle quali ogni cittadino possa ritrovarsi. Da questi obiettivi deriva la necessità di rivisitare il corredo di norme che regolamentano il terzo settore. È noto come la riforma del terzo settore adottata nel 2017 attendeva di essere completamente attuata. Proprio con questo provvedimento si coniuga l'interesse delle organizzazioni che ne fanno parte e che da anni aspettano delle risposte concrete nell'incertezza della piena entrata in vigore di tutte quelle disposizioni agevolative, ma anche per il sostegno alle importanti attività che queste associazioni quotidianamente svolgono nell'interesse della collettività, soprattutto a vantaggio dei più fragili. È davvero un provvedimento importante, colleghi, perché interviene su una materia delicata, a partire dagli assistenti sociali, donne e uomini che aiutano altre persone. A tal proposito sottolineo la deroga che supera i vincoli per le assunzioni degli assistenti sociali e nelle forme associative comunali per rendere sempre più capillare una presenza fondamentale nel territorio e rispondere a un fabbisogno che cresce e si modifica nel tempo. Questa deroga però al tempo stesso salvaguarda il rigore della gestione delle risorse finanziarie. Infatti le assunzioni possono avvenire nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale già esistenti e devono essere finanziate attraverso le risorse attualmente disponibili nei Fondi povertà e solidarietà comunale. Altra questione fondamentale che viene affrontata è quella che attiene all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori più vulnerabili. Viene istituito un tavolo di lavoro nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale dedicato ai minori che si trovano fuori dal contesto familiare, a coloro ai quali vengono affidati, ai servizi sociali territoriali e ai neomaggiorenni che si trovano in una condizione di prosieguo amministrativo. Con l'approccio coordinato e la messa a punto del sistema informativo si prevede pertanto un miglioramento significativo nella gestione delle informazioni riguardanti i minori affidati ai servizi sociali, finalizzato ad ottenere interventi mirati ed efficaci. Ricordo poi con soddisfazione che nella data del 9 aprile sarà istituita la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. Non si tratta di una delle tante giornate dedicate a un tema; certo, non risolve tutti i problemi, ma è davvero necessario ascoltare i minorenni anche nella sede giudiziaria. Si tratta quindi di un significativo segnale; uno strumento da affiancare a tante altre iniziative per tutelare la salute e il benessere psicologico dei minorenni, e che sarà utile a potenziare gli strumenti di ascolto. Altra novità riguarda le associazioni d'Arma. Con le associazioni nazionali dei Carabinieri o degli Alpini, sarà finalmente possibile iscriversi al ruolo unico nazionale del terzo settore per poter svolgere il loro prezioso lavoro, da sempre a vantaggio delle comunità e della protezione del bene comune, avvantaggiandosi del regime giuridico degli enti del terzo settore. Per queste ragioni, colleghi, e per molte altre, il provvedimento che ci apprestiamo a votare deve essere considerato un atto che farà la differenza per molte persone. È il segno di un'Italia ispirata dai suoi migliori valori solidaristici e che non vuole lasciare solo nessuno. Pertanto annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Con grande orgoglio ricordo una persona della mia terra scomparsa quarant'anni fa: il senatore Antonio Bisaglia, detto Toni Bisaglia. Ieri lo abbiamo ricordato in una commemorazione, con la Santa Messa; era anche presente il senatore Casini. Chi era Antonio Bisaglia e perché

rappresentare un territorio come il Polesine; l'ha saputo rappresentare per molti anni, rivestendo ruoli importanti, dal 1963 fino alla sua tragica fine, avvenuta quarant'anni fa, ieri, il 24 giugno 1984. È stato Ministro dell'industria, dell'artigianato e del commercio, è stato Ministro delle attività produttive, è stato Ministro dell'agricoltura, è stato Sottosegretario di Stato e nel suo ultimo incarico da deputato, poi passato per ininterrotti anni, dal 1963 al 1979, diventando senatore e presidente del Gruppo della Democrazia Cristiana in Senato.

non è facile a distanza di molti anni non tanto trovare memoria in una commemorazione, come a volte si fa in quest'Aula così importante, ma non è facile trovare un uomo come Antonio Bisaglia ancora nella memoria della gente di un territorio, che viene ricordato, che si è incarnato nel tessuto sociale di un territorio quale il Polesine. La sua tragica fine, discutibile e ancora incerta, è avvenuta quel 24 giugno 1984, in un tragico incidente, scivolando dalla barca morendo. Il fratello dedicò ulteriori dieci anni della sua vita per capire quali fossero le ragioni che determinarono la fine di Toni Bisaglia. Lo stesso fratello trovò fine poi nel lago

portando le istanze della propria terra e dell'intero territorio nazionale. Voglio ancora ricordarlo, per quanto ha fatto per noi e per dire a questa persona, che da quarant'anni non c'è più e che forse mi ascolta: grazie Toni, per quello che hai fatto per l'Italia, per il nostro Paese e per il Polesine.

avevo parlato in un intervento di fine seduta sei giorni fa, il 19 giugno, mercoledì scorso, di fronte a un'Aula svuotata, più o meno come quella di oggi. Evidentemente in quel caso un po' poco interessata al caso, che non era diventato ancora mediatico. Una macchina avvolgi-cavi gli aveva tranciato un braccio e provocato gravissime lesioni alle gambe e alla testa. Il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, anziché portarlo in ospedale, lo aveva abbandonato davanti alla sua abitazione gettando il braccio in una cassetta della frutta. Satnam non aveva il permesso di soggiorno, non aveva un contratto, veniva pagato pochi euro al giorno, così come migliaia di altri immigrati che lavorano nei campi e nelle fabbriche del nostro Paese. Oggi è a tutti evidente la drammaticità della vicenda, aggravata, se possibile, dal fatto che il padre del titolare dell'azienda, Renzo Lovato, a seguito dell'incidente aveva scaricato tutta la responsabilità dell'accaduto sul povero lavoratore indiano, colpevole secondo lui di non avere rispettato le indicazioni. Lo stesso Renzo Lovato risulta già da cinque anni indagato per caporalato dalla procura di Latina, che ha accertato i reati commessi tra il 2019 e 2020: indagini che dallo scorso luglio riposano tra i corridoi del tribunale tra cavilli, lungaggini burocratiche e difetti di notifica; colpevolmente, perché ancora non è stata fissata un'udienza preliminare. In questi giorni il Governo, per tramite della ministra del lavoro Calderone, ha annunciato più controlli e più ispettori. In questi due anni abbiamo perso il conto di quante volte siano stati fatti questi proclami, poi risolti nel nulla. È troppo tardi ora, anche rispetto alle parole pronunciate dal ministro Lollobrigida, che ha in qualche modo minimizzato il problema, parlando parlando di un incidente, come di un caso isolato. Purtroppo, Presidente, le morti sul lavoro sono aumentate e, invece che minimizzare, la politica e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Le leggi ci sono. Il Governo Renzi, con la legge che aveva voluto la ministra Teresa Bellanova nel 2020, aveva dato un forte impegno per cercare di contrastare lo sfruttamento e il caporalato, ma queste misure per funzionare devono essere finalizzate e applicate con vigore, hanno bisogno di finanziamenti costanti. Io penso che più che proclami, più che azioni comunicative, più che il tentativo come sempre di minimizzare si sia di fronte all'esigenza di una discussione vera Noi l'abbiamo chiesta, l'abbiamo chiesta nella Conferenza dei Capigruppo, l'abbiamo chiesta sin dal primo momento; ci è sembrato, anziché metterci a fare polemica, che il contributo giusto fosse aprire una riflessione seria su questo tema. Tra l'altro, qualche giorno dopo anche un altro ragazzo, Pierpaolo Baldini. di diciotto anni, è morto sul lavoro, in questo caso schiacciato da una macchina nella provincia di Lodi. Signora Presidente, conosco la sua sensibilità sul tema. La prego per cortesia di agire all'interno di tutte le sedi opportune, perché ci sia un confronto con i ministri Lollobrigida e Calderone quanto prima e che questo confronto possa essere un passo in avanti nel tentare almeno di individuare finanziamenti maggiori per i controlli e una discussione vera su come provare a evitare forme di sfruttamento così incivili, così gravi in quest'epoca moderna; cose che non dovrebbero nemmeno sentirsi in qualche modo e che purtroppo ancora ci sono. Io rimango stupefatta ancora una volta del fatto che parecchi colleghi hanno sentito di cosa stiamo parlando e siano usciti. È vero penso che non ci siamo proprio. Lo dico con sincerità e senza alcun intento di polemica. Però, di fronte a un tema come questo, anche cinque minuti alle ore 20 di sera forse possono valere

Senatrice Paita, questo è un tema che sta a cuore non solo a me e alla Presidenza, ma a tutta quest'Aula, che ha deciso di aprire proprio la seduta di oggi, se ricorda, con un minuto di silenzio in ricordo di

sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri che oscillano nella brezza del Sud, strani frutti che pendono dai pioppi». Era una canzone che riguardava ovviamente tempi che pensavamo abbandonati, quelli dello schiavismo; quelli in cui chi lavorava in quelle campagne e in quelle coltivazioni perdeva qualunque forma di dignità. Credo che dobbiamo essere tutti molto preoccupati del fatto che abbiamo visto scene che ricordano molto più quelle, che non quello che dovrebbe essere il lavoro ordinario, e forse dovremmo anche cambiare un po' il nostro linguaggio. Satman Singh non è morto per un infortunio sul lavoro: Satman Singh è morto perché, dopo un infortunio, è stato lasciato morire e si è deciso che doveva morire. Allora forse è più corretto chiamarlo omicidio che non infortunio sul lavoro. Ciò non toglie - lo ricordava il Presidente oggi pomeriggio aprendo la seduta - che Satman Singh è uno dei tanti nomi dei dieci giorni terribili che abbiamo alle spalle. Il Presidente non ha fatto in tempo a elencare un altro lavoratore che è morto oggi a Marghera, che, come Satnam Singh e come Diallo, fa parte di quei lavoratori che sono spesso negli appalti e sotto caporale. E allora spesso chiediamo, giustamente e necessariamente, che vengano i Ministri a riferire in Aula. Ne parliamo come necessità in un dibattito serio di quest'Aula su quei temi. Ma vorrei dire che abbiamo un grande problema:

Abbiamo anche un altro problema, e lo risottolineo: credo sia una vergogna che la Rai abbia aperto un servizio dicendo che si è trattato di una leggerezza del lavoratore di fronte a quello che si è dimostrato assolutamente un omicidio e - devo dire

di fare ciò che normalmente si farebbe (prestare soccorso e mettere in sicurezza il lavoratore) e perché si usano e si utilizzano i caporali. Credo allora che il messaggio che forse dobbiamo dare dare è che ci vogliono gli ispettori e l'applicazione delle leggi, però non possiamo continuare a raccontarci sempre gli stessi 800 ispettori: sono ventuno mesi che raccontiamo degli ispettori che erano stati decisi dal Governo Draghi. Forse la cosa che davvero dovrebbero fare i Ministri è - da un lato fare un nuovo concorso immediato perché ci siano davvero più ispettori e - dall'altro - mettere in atto le misure che la stessa legge sul caporalato prevede. Basterebbe che si dessero i dati sulla congruità perché un po' di caporali cominciassero a scomparire dalle nostre terre.

ha finalmente cancellato e tolto l'ambiguità tra l'attività produttiva e il diritto alla salute e all'ambiente di Taranto. Si tratta di una sentenza che, in maniera inequivocabile, evidenzia l'incompatibilità dell'impianto siderurgico con il diritto alla salute e all'ambiente. Oggi quella sentenza boccia anche il piano del Governo, Governo, che prevede un riutilizzo degli altiforni ormai quasi tutti spenti con l'utilizzo della tecnologia a carbone, chiaramente incompatibile non

certifica, sì, che c'è stata una riduzione del rischio di mortalità a seguito degli interventi programmati e realizzati all'interno dell'impianto, ma non sono stati assolutamente azzerati il rischio di mortalità

adotti tutte le misure per realizzare concretamente la riconversione economica, sociale e culturale del territorio e ponga fine al calvario degli oltre 7.000 lavoratori in cassa integrazione.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

Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 **(mercoledì 26, mattina)** - Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 **(mercoledì